Onorevoli Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri mattina, ha approvato a maggioranza il nuovo calendario dei lavori fino al 10 giugno. Nel corso di questa settimana - per la quale resta invariato il calendario già vigente - sarà discusso il decreto-legge sulla sospensione temporanea di demolizioni in Campania e proseguirà l'esame del disegno di legge di riforma della professione forense. Nella seduta pomeridiana di domani si svolgeranno - con trasmissione diretta televisiva - interrogazioni a risposta immediata al Ministro del lavoro sulla cassa integrazione guadagni. La prossima settimana, nelle sedute pomeridiana di lunedì 31 maggio e antimeridiana di martedì 1° giugno, sarà discusso il disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche, già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 19 di venerdì 28 maggio. Nelle sedute comprese tra l'8 e il 10 giugno, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche, sarà discusso il decreto-legge concernente spettacolo e attività culturali, per il quale sono stati ripartiti i tempi di esame.

i Gruppi della maggioranza e tutti i Gruppi dell'opposizione in ordine alla calendarizzazione del provvedimento sulle intercettazioni telefoniche a partire da lunedì prossimo. Il voto sul calendario è stato quindi un voto a maggioranza, come lei ha correttamente poc'anzi ricordato. Noi chiediamo che il calendario venga votato di nuovo in Aula su una proposta che io faccio,

Come i colleghi sanno, il provvedimento sulle intercettazioni telefoniche, già approvato alla Camera, arriva molti mesi or sono (credo ormai potremmo datarlo ad oltre un anno) al Senato. Per molto tempo non viene discusso; ne comincia poi la discussione in Commissione giustizia. Il testo che arriva è assolutamente insoddisfacente per l'opposizione. tuttavia solo l'opposizione che a questo testo muove delle critiche: è il più vasto mondo che riguarda l'informazione, gli editori, i magistrati (e in particolare la magistratura antimafia), moltissimi costituzionalisti, che si sono più volte espressi, e un'opinione pubblica allarmata. Il testo al Senato, nel corso della discussione (che è lunga e anche molto faticosa), viene ulteriormente peggiorato. Vengono introdotte limitazioni che impediscono chiaramente di poter avere notizia delle indagini a carico di qualunque soggetto, anche quando si tratti di fatti molto gravi (fatti di mafia, di terrorismo o che riguardino l'esercizio dei pubblici poteri o la gestione delle pubbliche risorse) per anni e anni: un vero sistema di censura. Dall'altra parte, vengono limitati gli ambiti della possibilità di utilizzo delle intercettazioni, non solo telefoniche, ma anche ambientali e telematiche, da parte della magistratura inquirente, con limitazioni che riguardano i tempi, ma anche le occasioni e i momenti in cui tali intercettazioni possono essere compiute. Unica novità positiva è la modificazione di uno dei presupposti per l'ammissibilità delle intercettazioni, che è quello che riguarda la sostituzione della espressione «elementi di colpevolezza» con l'espressione «gravi indizi di reato». Ma l'attività di peggioramento del testo, affidata da una parte al relatore di maggioranza e dall'altra parte al consenziente - sempre consenziente - rappresentante del Governo, procede inesausta. Eppure, è materia sulla quale benissimo opposizione e maggioranza avrebbero potuto trovare un punto d'incontro. Infatti, che si debba riformare la materia delle intercettazioni per una più accurata e seria tutela della *privacy* dei soggetti e della dignità di tutti coloro i quali vengono intercettati, qualunque sia lo strumento delle intercettazioni, essendo estranei alle indagini, o per limitare la diffusione di notizie che riguardino la vita privata o aspetti non inerenti alle indagini, sia di estranei alle indagini stesse, sia degli stessi indagati, stessi indagati, è un'opinione talmente condivisa in questo Parlamento che già dalla scorsa legislatura si sono succeduti disegni di legge, alcuni dei quali provenienti non soltanto dal Governo, ma anche da questo Gruppo. Voglio ricordare quelli presentati in questa legislatura: uno come primo firmatario ha il senatore Casson e

molto facilmente trovare un accordo. Ma evidentemente lo spirito non era questo, e l'attività indefessa di peggioramento del testo operata dal relatore di maggioranza e dal rappresentante del Governo, evidentemente in esecuzione di un *input* politico netto (direi anche nettissimo) continua senza sosta. I numerosissimi emendamenti presentati dalle opposizioni, tutti minuziosamente illustrati (e non per fare ostruzionismo, come ieri ha ricordato lo stesso presidente Berselli in una lettera che, peraltro, ha aspetti che non condivido, su cui tornerò molto brevemente dopo), danno atto all'opposizione di aver tentato di migliorare questo testo e di ricondurlo nell'alveo di quello che avrebbe dovuto essere, e cioè un provvedimento serio a tutela della *privacy* e del segreto istruttorio.

straccia, poiché una modifica seria, invadente - immagino - dello stesso è già pronta per essere presentata dal Governo. Noi ci troveremo, quindi, nella bizzarra situazione in cui, dopo aver impiegato

drammatica finzione che si aggiunge alla mistificazione di un testo che avrebbe dovuto tutelare la *privacy* e il segreto istruttorio e che in realtà serve a limare le unghie ai magistrati e ad instaurare la censura in questo Paese. La chiamo così com'è: la censura. lei capisce che l'opposizione non può lasciar fare. Io mi stupisco che lascino fare i senatori della maggioranza. Da ieri si susseguono dichiarazioni di rappresentanti del centrodestra della Camera, i quali dicono che il testo verrà cambiato, che si tornerà al testo della Camera, che grandi modifiche verranno fatte. Non voglio pensare alla mortificazione del rappresentante del Governo e del relatore di maggioranza che con tanta forza, talvolta ottusa - lasciatemelo dire - e sorda alle richieste dell'opposizione, hanno continuato a perseverare nel peggioramento ulteriore di questo drammatico testo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Ma mi riferisco, colleghi, anche all'autorevolezza di questo Senato. all'autorevolezza di questo Senato. E per non essere offensiva farò un paragone che coinvolge, avvocato Longo, non soltanto i senatori della maggioranza, ma anche quelli dell'opposizione: ci troviamo nella straordinaria situazione nella quale si trovarono quei soggetti che accompagnavano i muli sui quali venivano caricate le vettovaglie e gli armamenti nella Prima guerra mondiale, chiamati a scalare montagne pietrose e pericolose per poi magari sentirsi dire che c'era un contrordine: per che diavolo di motivo avevano fatto la fatica di salire su? Che scendessero in pianura, dove gli ufficiali, splendenti nelle loro divise, andavano con la vittoria scritta in fronte verso la battaglia. Francamente, credo che né i senatori della maggioranza, né i senatori dell'opposizione, né il Senato in quanto tale possano sopportare l'oltraggio di farsi dettare a che cosa dire «signorsì»!

Non siamo disponibili a farci imporre da nessuno un testo: e questo lo dico in un momento in cui, tra l'altro, mi si lasci dire, non vedo l'urgenza, la straordinaria urgenza di questo provvedimento. Ieri abbiamo approvato il provvedimento sulla Grecia e abbiamo chiesto che il ministro Tremonti venga in Aula, in un clima di amicizia, Presidente e colleghi, non in un clima di ostilità, per spiegarci qual è la situazione europea, perché ci apprestiamo ad esaminare una manovra - che voi dite essere di 24 miliardi di euro, ma in realtà è di 36 miliardi - che imporrà lacrime e sangue all'Italia e soprattutto ad alcuni soggetti, come sempre quelli più esposti, quelli più facilmente raggiungibili. questo arde, mentre i giornali di tutto il mondo portano in prima pagina le notizie che riguardano la crisi europea, noi dobbiamo romperci il collo per affrontare un testo non sapendo di che cosa stiamo parlando! Credo che questo sia inaccettabile perché noi sappiamo bene di cosa stiamo parlando: stiamo parlando della libertà di informazione, del diritto dei cittadini di sapere

le parole della presidente Finocchiaro ci fanno venire in mente l'immagine di un Senato di fatto commissariato. Un Senato commissariato possiamo scegliere da chi: se dal Presidente del Consiglio, dai suoi consiglieri giuridici, dal Presidente della Camera. Di fatto questa Camera, presieduta dalla seconda carica dello Stato, è comunque commissariata e, quindi, incapace di decidere autonomamente. Questa è un'offesa incredibile, ma soprattutto ci sembra una riscrittura apocrifa della nostra Costituzione. In questi giorni ne abbiamo viste di tutti i colori,

quei mentecatti presenti in Commissione - e tra questi c'ero anch'io in quel momento - stavano perdendo il loro tempo perché si stava per cambiare il testo. È evidente che questo è l'ennesimo strappo fatto in un momento particolare del Paese, probabilmente per mettere una pietra tombale su "criccopoli", probabilmente per nascondere il letamaio che sta venendo a galla nella gestione della Protezione civile, probabilmente perché nulla si deve sapere nel momento in cui un Governo che aveva detto che l'Italia era il Paese di bengodi poi fa manovre che lo ridurranno ancora di più con le pezze al sedere. Quindi, Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori, che pure ha lavorato tenacemente in Commissione, con il collega Li Gotti che, puntualmente e senza tecniche ostruzionistiche, è entrato nel merito dei singoli articoli e delle singole misure,

al netto dei toni elegantemente enfatici che sono naturali, anzi doverosi per il capo dell'opposizione in un ramo del Parlamento, condivido pienamente l'intervento della presidente Finocchiaro.

È vero che questo provvedimento è da molto tempo all'attenzione dell'opinione pubblica, accompagnato anche da giudizi fortemente divergenti, che segnalano un interesse profondo profondo attorno a questa vicenda, ma esso è stato oggetto di un impegno della Commissione parlamentare del Senato all'indomani

carico di un ulteriore "avanzamento" in termini restrittivi di questo testo, che ha incontrato forti critiche, è vero, non nella magistratura associata (poteva essere una classica *querelle* tra giustizia e politica),

ogni giorno di più è avanzata la critica nel campo dell'informazione, dell'editoria, di un sistema che avverte questo provvedimento come pericolosamente lesivo del diritto di informazione,

provvedimenti fortemente modificativi di questo testo, che dovrebbero riportarne la formulazione a quella varata dalla Camera dei deputati qualche mese fa,

ma misurando la propria scelta in ragione del testo presentato, aspettano di comprenderne il contenuto per decidere come votare? Abbiamo già preannunciato, signor Presidente, che se il testo sarà quello

Ma se il testo sarà profondamente diverso, allora la posizione si misurerà con il contenuto dello stesso. Non le pare, anche per quanto ci riguarda, del tutto improprio costringerci alla valutazione di un testo superato? assolutamente incongruo che la maggioranza debba difendere un testo che è già altro?

per una riflessione più approfondita sulle intercettazioni che permetta il dispiego pieno della manovra finanziaria. Credo che la ragionevolezza e la volontà di preservare un sistema di relazioni politiche in termini istituzionali, ma anche all'interno di aree politiche che possono non essere contrarie consiglierebbero alla maggioranza parlamentare qui, al Senato, di recedere da questa proposta di calendario.

si dovesse passare all'esame di altre problematiche sicuramente più importanti per il Paese, come la crisi economica. Quindi, ci aspettavamo che nella calendarizzazione

non fosse altro perché questa manovra finanziaria così importante incide sicuramente sulla nostra economia, ma anche sui bilanci di tante famiglie italiane. E siccome sappiamo che saranno tanti i sacrifici che andremo a chiedere

Al contrario, insistiamo sulle intercettazioni telefoniche dimenticandoci, tra l'altro, che abbiamo accantonato un disegno di legge sulla riforma della professione forense, che

Avevamo apprezzato la possibilità che la maggioranza aveva espresso di un confronto reale anche sulle intercettazioni telefoniche:

Il buonsenso, se così possiamo chiamarlo, avrebbe voluto che, come prima emergenza, fosse aperta una sessione di bilancio, con un approfondito esame della manovra finanziaria,

Nel frattempo, si sarebbe potuto lavorare anche sul disegno di legge sulle intercettazioni per sciogliere quei nodi che, come sappiamo tutti, esistono e devono essere affrontati se vogliamo una legge che sia oggettivamente condivisa da tutti.

di molte strumentalizzazioni e di una buona dose di populismo, anche mediatico, su un tema che sappiamo tutti essere molto delicato.

fascista del 1930 non poneva alcun limite alle intercettazioni, che potevano essere effettuate per qualsiasi tipo di reato, senza un termine di durata e senza nessun tipo di verifica sui presupposti del provvedimento autorizzativo.

da molti esponenti della sinistra e se possiamo capire che l'ideologia fascista possa attrarre una parte minoritaria della maggioranza che ad essa si rifaceva, non riusciamo a capire come possano diversi esponenti del centrosinistra sostenere una posizione analoga a quella del codice del 1930, che prevedeva di lasciare liberi i magistrati di procedere con questo strumento investigativo senza alcuna limitazione. Su questo tema si sono misurati tutti i Governi, anche il Governo Prodi con il ministro Mastella, e ho sentito dire che bisogna tornare al loro testo. Andate a vedere che cosa dice quel testo sul regime di pubblicabilità degli atti di indagine: a mio avviso è molto più rigoroso di quello che abbiamo proposto noi e che ha proposto il Governo attuale, che si sta ora analizzando e che verrà esaminato dall'Aula.

per quanto sia difficile - e lo sanno i colleghi della sinistra trovare una soluzione equilibra su un tema su cui scontrano quattro valori costituzionali completamente opposti:

confliggono tra loro e trovare una soluzione non è semplice, prova ne sia che Prodi e Mastella, dopo aver proposto un testo che venne approvato dalla Camera senza nessun voto contrario, dovettero abbandonare la loro idea di riformare questo settore. Ho sentito dire prima dalla presidente Finocchiaro, le cui opinioni ascoltiamo sempre con attenzione, che il testo della Camera è migliore di quello uscito dalla Commissione giustizia del Senato.

chiediamo come presupposto di ammissibilità di questo strumento investigativo, così efficace ma così insidioso, che sia necessario avere un quadro indiziario di colpevolezza della persona intercettata per procedere all'utilizzo di tale strumento?

perché è chiaro che il pubblico ministero ha interesse ad usare questo strumento anche per iniziare le indagini e non per proseguirle, come dice il codice attuale,

per rivedere questa norma che fa riferimento all'articolo 684 del codice penale che sanziona la violazione della segretezza investigativa, fattispecie di reato per la quale, in verità, in Italia non è mai stato condannato nessuno. Quindi, sappiamo che sono anche sanzioni molto virtuali, che non sono mai state applicate e probabilmente non lo saranno mai. Ma le sanzioni hanno anche un valore simbolico.

non sarà un equilibrio perfetto, anche perché su questo tema non esiste l'equilibrio perfetto ma solo un contemperamento di esigenze. Riteniamo che quel testo che la Commissione giustizia ha prodotto, sia un testo che cerca di trovare un equilibrio, anche se siamo disposti a rivederlo in alcuni passaggi. Sia chiaro però che su questo *iter* legislativo bisogna arrivare alla conclusione, cercando di incidere il meno possibile sulla libertà delle persone e dando ai magistrati, che hanno l'obbligo di essere professionalmente preparati, l'uso di uno strumento investigativo e non l'abuso, com'è stato fino ad oggi. Signor Presidente, la maggioranza e il Gruppo PdL sono assolutamente consapevoli della delicatezza della materia che fa riferimento alle intercettazioni. Sappiamo, e lo sapevamo dall'inizio, che sono in discussione in questo provvedimento esigenze legittime e contrapposte, che meritano tutte tutela e che devono essere armonizzate cercando un punto di equilibrio e un punto di caduta. Sono, peraltro, tutte esigenze protette costituzionalmente. Vi è da una parte l'esigenza delle indagini, innanzitutto nei confronti della criminalità organizzata.

parte, c'è l'esigenza di tutelare un margine di riservatezza per tutti i cittadini.

debba essere considerato a geometria variabile. Credo però che ci troveremmo in un Paese incivile se non garantissimo anche all'ultimo dei cittadini o anche a quello più esposto pubblicamente un margine di vita privata. Abbiamo tutti visto un bellissimo film sulla Germania orientale, dal titolo «Le vite degli altri», che evidenziava quanto e fino a che punto, attraverso un sistema di intercettazioni, che tra le altre cose non sfruttava nemmeno nemmeno le ultime innovazioni della tecnologia, si potesse devastare la vita dei comuni cittadini. Quel film ha prodotto emozione persino in quanti, signor Presidente, provengono da quella tradizione comunista

signor Presidente, un punto di caduta e di mediazione si deve tra un sacrosanto diritto di cronaca e diritti che esistono anche in capo all'imputato,

di ciò di cui si risponde di fronte alla giustizia. E questa esigenza è bene che sia tutelata dal giudice naturale, non da fughe di notizie che appaiono il giorno dopo sui quotidiani e che magari sono state causate dal fatto che i fascicoli sono stati abbandonati sulla scrivania con la porta aperta

che, nella mediazione tra queste esigenze, che nessuno nega, vi siano punti di vista differenti tra la maggioranza e l'opposizione. In caso contrario non saremmo all'interno di un sistema democratico, non saremmo all'interno di un sistema parlamentare. Questa è una di quelle materie che fa venire a galla le esigenze di fondo che sono a cuore a schieramenti che nell'emiciclo si trovano in posizione contrapposta. Una volta acclarato questo Una volta acclarato questo dato, e consentito alla maggioranza di pensarla in modo diverso dall'opposizione, è necessario però riflettere, pensare, ponderare le decisioni, soprattutto nel momento in cui vi sono esigenze così importanti in discussione. Vorrei ricordare brevemente

Questo vuol dire che, alla prova della coscienza, tradotto in termini secolari, alcuni membri dell'opposizione hanno votato con la maggioranza. Quel testo è stato approvato ed è approdato in discussione in Senato, in Commissione. La Commissione ha preso innanzitutto in considerazione l'ipotesi di fare un passo indietro su un aspetto importante che faceva riferimento alle indagini, proprio perché evidentemente era interessata a fare le indagini potessero ricevere il minore nocumento possibile dalla garanzia dei diritti personali. Ritengo, senatrice Finocchiaro, che siamo tutti d'accordo sul fatto

contrarietà esplicita dell'opposizione, come è normale che sia, ma anche di alcune voci all'interno del Paese. Di fronte a questa situazione, la maggioranza ha affermato che avrebbe lasciato il testo aperto anche in Aula, evitando di blindare un provvedimento che pure è stato il frutto di un anno di lavoro e di scontro in Commissione. Tutti sanno, perché hanno esperienza parlamentare, che esistono strumenti

a nome del mio Gruppo sono in grado di dare due assicurazioni alla senatrice Finocchiaro. La prima è che il lavoro della Commissione non è lavoro che andrà vanificato ed è lavoro di cui si terrà conto e di cui resterà traccia profonda nel provvedimento finale. Le seconda è che nessuno intende acquisire qui, come se fossimo dei semplici operatori, dei semplici

che è stata indicata, li firmeremo e li discuteremo in un pubblico confronto con l'opposizione. È questo quello che ci chiede il parlamentarismo. Stiamo vivendo un momento che esalta il parlamentarismo.

non arriveremo in Aula con situazioni sfilacciate, anche per darvi la possibilità di contrastarci meglio. Lo facciamo anche per rispetto della vostra funzione.

La mia richiesta riguarda la revoca del contingentamento dei tempi assegnati all'Assemblea per la discussione di questa materia. Veniamo da due settimane di sedute di Commissione giustizia, ripetute a ritmo incalzante: sedute anche notturne. È stato un lavoro caratterizzato da una pressione temporale e da una fretta eccessive e incomprensibili in una logica istituzionale corretta. La fretta, inconsulta e inopinata, è stata da noi fortemente contestata, soprattutto nel corso delle ultime sedute, durante le quali peraltro ci siamo resi conto dell'assoluta inutilità del nostro lavoro e durante le quali abbiamo assistito a sonore dormite notturne da parte di senatori della maggioranza: una situazione quasi kafkiana, del tutto assurda. Di fronte ad un Ministro della giustizia che pubblicamente, davanti alla stampa, sconfessava la sua maggioranza, compreso il relatore di maggioranza, affermando che alcune modifiche apportate al testo pervenuto dalla Camera dei deputati erano iniziativa di singoli senatori della maggioranza e non del Governo, si è creata una situazione paradossale. Abbiamo ora un testo del disegno di legge Alfano approvato in Commissione già sconfessato dallo stesso Ministro; non sappiamo quale sarà il testo reale, il vero testo del disegno di legge Alfano. Stiamo discutendo, tra Camera e Senato, tra Commissioni di merito e Commissione antimafia, di nuove norme in materia di criminalità organizzata, di lotta alla mafia, di lotta alle ecomafie, di prevenzione e lotta alla corruzione, tutte norme che in un modo anche diretto avranno a che fare con il disegno di legge sulle intercettazioni, perché da una parte Governo e maggioranza parlano di sicurezza e di lotta alla criminalità come priorità, dall'altra parte Governo e maggioranza impediscono alla polizia di lavorare, limitano i mezzi investigativi come le intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali. Allora, per salvare Governo e maggioranza da una incipiente schizofrenia istituzionale, li invitiamo a schiarirsi le idee, a prendere decisioni adeguate e coerenti. Concretamente cosa significa tutto ciò? Dovrebbe significare che in questa Aula del Senato dovremmo conoscere per tempo il nuovo testo del disegno di legge; dovremmo avere il tempo adeguato per discutere, preferibilmente in Commissione, ma anche in quest'Aula, delle norme in una materia così complessa e delicata; dovremmo studiare gli emendamenti da proporre. Chiediamo quindi che da parte dell'Assemblea si disponga la revoca del provvedimento di contingentamento dei tempi di discussione in quest'Aula. Riteniamo che un'ora, un'ora e mezza circa di tempo riservata ai 114 senatori del Partito Democratico sia veramente offensiva, un'offesa alla dignità non solo dei singoli senatori, ma della stessa istituzione parlamentare. Con il disegno di legge Alfano sulle intercettazioni già avete dimostrato di voler mettere le manette alla polizia, di voler mettere il bavaglio alla stampa. Evitate almeno ora di imbavagliare il Parlamento; evitate di imbavagliare il Senato!

La premessa è che davvero mai mi sarei immaginato, prima di questa esperienza parlamentare e durante questa esperienza, di dover assistere ad una vera e propria operazione di introduzione della censura nel nostro Paese, perché le parole sono quelle che servono per definire le situazioni. Siamo di fronte ad un disegno di legge, quello della cui calendarizzazione oggi ci accingiamo a discutere, che riesce ad ottenere un triplice risultato, che esemplificherei con le reazioni dei futuri potenziali protagonisti. Immaginiamo che cosa pensano - non è difficile immaginarlo, basta parlarci - gli appartenenti alle forze di polizia e ai reparti investigativi dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza di fronte a questa legge: sono sgomenti. Immaginiamo che cosa pensano i giornalisti, quale che sia la loro collocazione politica e ideologica, di fronte a questa legge: sono sgomenti. Immaginiamo che cosa pensano di fronte a questa legge i criminali: credete che siano sgomenti? No, sono molto contenti dell'arrivo di questa legge. *(Applausi dal tre categorie di soggetti: poliziotti, carabinieri e finanzieri da un lato e giornalisti dall'altro, che attendono sgomenti l'arrivo di una legge censura che paralizza l'attività di indagine; e poi ci sono i criminali che si accingono

del singolare e surreale percorso in Commissione, assistiamo oggi alle irrituali promesse di totale modifica del testo del testo formulate nell'anticamera della Commissione giustizia dal Guardasigilli. Sono pertanto qui a richiedere, perlomeno a modifica del calendario a suo tempo fissato, una dilazione di tre settimane, per consentire uno studio e un approfondimento adeguati del quadro normativo definito dal disegno di legge approvato in Commissione e da quello, probabilmente del tutto diverso, che viene in qualche modo prospettato - temo in peggio, visto che il percorso di questo disegno di legge è tutto in discesa verso il baratro del disastro istituzionale - per consentirci almeno di esaminarlo

mia proposta di modifica del calendario prevede di dedicare la giornata di lunedì e martedì ad un dibattito sulla situazione economica alla presenza del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'econimia: dobbiamo chiederci quale sia in questo momento l'urgenza assoluta nell'agenda del Parlamento. Io penso che sia la situazione economica: le parole

Le parole e il richiamo preoccupato e responsabile del presidente Napolitano indicano pur esse una situazione di particolarissima gravità della situazione economica del nostro Paese. Ora, di fronte a questa situazione, qual è il compito dell'opposizione? Io penso non debba essere quello di limitarsi a sfruttare in modo più o meno demagogico le difficoltà. Potremmo limitarci a dire, come ho ricordato ieri, che in questi ultimi due anni la spesa pubblica in Italia è cresciuta di 51 miliardi e che se il Governo in carica avesse mantenuto la buona eredità eredità del Governo precedente oggi non si richiederebbe una misura così pesante per la situazione dei conti pubblici; ma è chiaro che ben sappiamo che ci sono dei problemi strutturali nel Paese e dunque, ove chiamati ad una responsabilità, saremo pronti a dare il nostro contributo e ad esprimere le nostre posizioni su ciò che in questo momento serve al Paese. è un compito dell'opposizione e naturalmente vi è anche un dovere della maggioranza. Se la situazione è così grave come è stata descritta, c'è un dovere precipuo della maggioranza a cui gli italiani hanno affidato il compito di governare: penso che sia quello di concentrarsi sulla priorità assoluta, su questa manovra così impegnativa, sgombrando il campo da tutto ciò che può dividere il Paese. Questa ostinazione nel portare avanti come priorità assoluta una una proposta che sta dividendo il Paese non solo tra maggioranza e opposizione, ma che vede all'opposizione tutta l'area delle forze che lo Stato mette in campo per combattere la criminalità

perché sia possibile un incontro sulle cose sostanziali e su questa emergenza. E allora c'è una premessa, signor Presidente: magari poi sulle soluzioni tecniche potremo anche dividerci, dovremo cercare di costruire le condizioni di una convergenza nell'analisi e nell'individuazione delle priorità. Lo abbiamo detto ieri e lo ripeto oggi. Per queste ragioni riterrei preliminare all'esame di merito della manovra una grande discussione politica che segni una presa di coscienza collettiva sulla reale situazione economico-finanziaria del nostro Paese. Signor Presidente, alcuni colleghi nel corso di questi giorni hanno

È mia opinione - e penso sia un'opinione condivisa da molti altri colleghi della maggioranza e dell'opposizione - che il tema sul quale noi ci siamo soffermati nelle 39 sedute della Commissione, comprendendo anche alcune audizioni, sia di estrema delicatezza e importanza. Non se ne parla dal 1930; ho colto le acute osservazioni del senatore Mazzatorta,

non possiamo riferirci al codice Rocco in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali, non fosse altro perché la scienza non era ancora approdata

Paese è iniziato nel 1997, da quando si cerca di intervenire per meglio regolamentare questa materia molto delicata.

che, su un testo composto da un unico articolo distribuito su 35 commi, la Commissione giustizia del Senato ha apportato 34 modifiche:

24 su suggerimenti emendativi del Governo e del relatore. Su un gran numero di altri punti - circa 20 le riflessioni emendative sono state respinte con un voto tecnico, ma con l'impegno da parte del Governo e della maggioranza di una loro considerazione per l'Aula. Non è un caso, Presidente, che il presidente Berselli abbia scritto a noi, componenti della Commissione, che l'Aula con il contributo di tutti saprà apportare quelle ulteriori modifiche migliorative di cui abbiamo ampiamente parlato: ossia, se ne è parlato. Questo Questo avveniva fino a lunedì mattina; da lunedì è cambiata la situazione. Pare che il testo non potrà essere più questo; ovviamente l'Assemblea, nella sua sovranità, potrà decidere, ma se dovesse configurarsi

Noi abbiamo veramente lavorato, in trentanove sedute, per cercare di offrire al Paese uno strumento utile, nell'interesse dei cittadini e della giustizia. Abbiamo fatto bene o male, siamo soddisfatti o non lo siamo, ma abbiamo lavorato. Non si può, da sedi esterne rispetto a quella nella quale noi abbiamo contribuito con il nostro lavoro, comunicare che il testo sarà diverso! Se sarà diverso lei, signor Presidente, tuteli il nostro lavoro,

delle posizioni. Anche quando si discute di poesia si può litigare, figuriamoci quando si discute di questi temi. Ma si tratta di un confronto sempre tecnico, le assicuro. Ne è buon testimone il lavoro svolto dal presidente Berselli, che ha riconosciuto il valore tecnico del confronto. Riassegni, qualora dovesse manifestarsi questo tipo di evoluzione,

tutte le manifestazioni che sono state fatte. Voi siete riusciti a ricompattare direttori di giornali di destra e di sinistra, da Vittorio Feltri a Ezio Mauro, a Ferruccio De Bortoli, perché temono che questa legge possa mettere un bavaglio all'informazione. Voglio solo portare alcune testimonianze. Nel 2005 alcuni immobiliaristi volevano scalare la Banca Antonveneta Antonveneta e il «Corriere della Sera»: senza le intercettazioni telefoniche quell'operazione sarebbe riuscita. Voglio ricordare

recupero a vantaggio del fisco e dei contribuenti di un'evasione fiscale. Voglio ricordare, e lo ricordo dal marzo dell'anno scorso, la questione della degli appalti: se non vi fossero state le intercettazioni telefoniche avrebbero continuato impunemente nel loro malaffare. Voglio ricordare, signor Presidente, un articolo di oggi sul quotidiano «la Repubblica»; Liana Milella, una bravissima giornalista che segue i nostri lavori, scrive, riportando parole del presidente del Consiglio Berlusconi: «Approviamo questa inutile legge al Senato e poi mettiamola su un binario morto. Ha già creato troppi problemi». Voglio ricordare un articolo dove il capo della Polizia Manganelli ha affermato che questa legge bavaglio mette gravemente a rischio la lotta alla mafia. Non voglio citare magistrati come Ingroia e come gli altri che indagano e ritengono che sia un dovere quello di intercettare per lottare contro il malaffare, contro la corruzione. Voglio ricordare altri

non avete alcun diritto di violare la Costituzione, le libertà dei cittadini e il diritto ad avere un'informazione libera, pluralistica. I giornalisti sono già attaccati: voglio ricordare - e termino, signor Presidente - che ci sono giornalisti con la schiena dritta, come Gatti de «L'espresso», ai quali vengono chiesti 26 milioni di euro di risarcimenti perché denunciano le disfunzioni delle Ferrovie dello Stato e la situazione di pendolari che viaggiano come merci. Concludo il mio intervento, pregando tutti quanti: per combattere la corruzione, come voi dite, non si può mettere il bavaglio all'informazione. Ritirate questa proposta di legge e ve ne saranno grati tutti gli italiani. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il contesto in cui ci troviamo a discutere produce un effetto involontariamente ironico. Se le notizie di stampa a proposito del tema di cui parlerò saranno confermate, abbiamo di fronte una situazione in cui lo stesso Presidente del Consiglio ha a suo tempo registrato ed intercettato i propri dipendenti, nelle proprie residenze, sottoponendo la platea delle persone che lavorano per lui ad una sorveglianza occhiuta e nascosta. In secondo luogo, se le notizie di stampa saranno confermate, come sta avvenendo, il Presidente del Consiglio ha potuto approfittare delle registrazioni che riguardavano alcuni esponenti dell'opposizione in conversazioni private ed ha potuto utilizzare queste intercettazioni per giocarle come materia prima bollente all'interno della campagna elettorale. Noi subiamo una situazione in cui il Presidente del Consiglio in persona ha lucrato su un uso illegittimo delle intercettazioni e dobbiamo subire una situazione in cui dalla maggioranza che ha espresso questo Presidente del Consiglio ci vengono proposte lezioni di riservatezza e di democrazia che chiudono il diritto all'informazione. Ci sono due aspetti importanti di questa faccenda e purtroppo negli ultimi tempi ci stiamo occupando soltanto del secondo. È l'importantissimo diritto all'informazione, come hanno detto illustri costituzionalisti come Onida e Pace: c'è il diritto ad essere informati e ad informare. Sono due diritti complementari che sorreggono la conoscenza, il diritto alla conoscenza da parte dei cittadini, senza di che non c'è nemmeno la possibilità di esprimere pareri ragionati nel dibattito democratico. C'è di fronte a noi un progetto di vera e propria omertà di Stato, perché si propone un meccanismo legislativo per cui i proprietari dei giornali, gli azionisti di maggioranza degli organi di stampa saranno invitati a far essi stessi i censori dei propri organi di stampa per evitare di dover subire delle condanne e delle multe di proporzioni bibliche. Ma c'è un altro aspetto che il dibattito giustissimo sulla libertà di stampa in questo momento sta mettendo a lato, ed è il fatto che c'è una parte di questa legge che "chiude" sostanzialmente l'uso delle intercettazioni, ne rende l'accettazione farraginosa, complicata, viscosa. Alla fine non avremo più le intercettazioni e allora non ci sarà più nemmeno il problema se i giornalisti avranno la possibilità di scriverne e pubblicarne, perché si cerca di chiudere all'origine questa fonte di informazione. Ora abbiamo davanti a noi questa situazione e, di fronte ad essa, una consapevolezza: ciò che noi abbiamo saputo negli ultimi anni dalle intercettazioni è stato prezioso per la formazione della coscienza collettiva e della conoscenza e del diritto alla conoscenza. Sapere che un Ministro si fa pagare la casa da un'altra persona

Ricordo ai colleghi di questo Gruppo che gli interventi devono essere finalizzati alla richiesta di modifica del calendario e, quindi, possono essere contenuti in uno spazio temporale che consenta al senatore di esprimere la propria richiesta e all'Aula di conoscere

Io voglio evitare qualunque forma di incidente. Consento a ciascun collega di parlare e di illustrare la propria richiesta di modifica del calendario. È in atto una forma di corretto ostruzionismo. Lungi da me l'idea di entrare nel merito. Voi esercitate i diritti previsti dal Regolamento. Anche la Presidenza, come voi sapete, è tenuta ad armonizzare i tempi per garantire il corretto andamento dei lavori. Quindi, bisogna trovare una sintesi. Questa Presidenza deve incardinare un provvedimento altrettanto urgente. Come ieri ha dato priorità ad una vostra richiesta altrettanto accettabile, quale quella della trattazione del decreto sulla oggi ritiene che, esaurita la fase dei vostri interventi, si debba dare altrettanta importanza ad un rilevante decreto che sospende le demolizioni in Campania. Quindi, chiedo anche al Gruppo del Partito Democratico un reciproco gesto di collaborazione, come quello posto

Presidente, noi non possiamo accettare la sua decisione, e non possiamo farlo perché è gravemente lesiva del diritto di ciascun senatore,

appunto, dal Regolamento, quella di proporre all'Assemblea di articolare i propri lavori in modo diverso da quanto la Conferenza dei Capigruppo maggioritariamente ha stabilito. È assolutamente vero che lei ha

non corrisponde ad un corretto esercizio di questo potere, discrezionale sì, ma che deve svolgersi entro limiti di ragionevolezza. Voglio ricordarle, signor Presidente, nella seduta del 14 novembre 2007 proprio su questo tema, ovvero sull'esercizio dei poteri del Presidente di armonizzare la discussione esattamente sulle proposte di modifica del calendario.

Ha una sua logica in presenza di una scadenza di decreti-legge, di norme che vanno approvate inderogabilmente entro una certa data, pena la loro decadenza». demolizioni in Campania ha appena iniziato il suo *iter* e non abbiamo altre scadenze imminenti ed immediate; non c'è alcuna ragione per comprimere questa fase della discussione. D'altra parte, signor Presidente, ieri, quando abbiamo formulato la la proposta di anticipare la discussione sul decreto Grecia, gli altri Gruppi hanno aderito, e lei ha disposto conformemente alla volontà espressa, proprio per avere il tempo - fu espressa tale volontà tale volontà - di articolare questa discussione e le successive votazioni, che, non ho bisogno di ricordarlo, rientreranno per ciascuna delle singole proposte di modifica del calendario entro i tempi necessari, né più né meno. Non c'è nessuna ragione per la quale del decreto Campania debba essere incardinato alle ore 13. Noi non ci sentiamo vincolati a questa indicazione, che non è recata nel calendario e non risponde a esigenze di scadenza improrogabile. Per questa ragione le chiediamo, riconoscendole ovviamente il potere di armonizzare nei termini che ho detto prima, di voler concedere almeno quattro minuti per ciascun componente del nostro Gruppo che voglia proporre una proposta alternativa di calendario. *(Applausi io ho degli illustri precedenti. Non è mia volontà arrivare ad un conflitto con le vostre richieste che vengono svolte in funzione dell'esercizio di un diritto regolamentare, ma si tratta di trovare un punto di buon senso. Io ho anche dei precedenti che vanno nel senso del contingentamento da un minuto fino a due o tre minuti. Vi sono precedenti che vanno in tutti i sensi; non trovo precedenti di armonizzazione con interventi di quattro minuti in presenza di notevoli richieste.

Ci sono dei precedenti. Se vuole, le cito un precedente del presidente Marini. Se volete arrivare necessariamente allo scontro con la Presidenza fatecelo sapere, noi siamo qui e lo accettiamo, però da parte di questa Presidenza si sta cercando di tutto per trovare un momento di sintesi.

Presidente, prendo la parola per dirle esattamente il contrario di quello che lei poco fa denunciava: noi non vogliamo lo scontro con la Presidenza e operiamo perché questo scontro non ci sia. Riteniamo che tale provvedimento sia di capitale importanza, e su ciò l'intero Gruppo del Partito Democratico concorda. Abbiamo la necessità di esprimere,

Ciascuno di noi ha bisogno, come lei comprende, di dare un minimo di argomento alla proposta di modifica del calendario. La ringrazio sin d'ora, aspettandomi che lei possa accedere a questa richiesta.

Marini stabilisce l'armonizzazione dei tempi per il prosieguo degli interventi: due minuti. Il presidente Marini disse: «Ora però, per illustrare le proposte, vi prego di impiegare solo uno o due minuti: non possiamo andare oltre, altrimenti salterebbe l'impegno di armonizzazione del Presidente. Vi prego di stare a questi tempi, di rispettarli, altrimenti non ci siamo». E si trovò l'intesa. Ero io Capogruppo di opposizione. E ancora: «Darò la parola soltanto per presentare richieste che non siano già contemplate dalle due formali avanzate dai senatori Schifani e D'Onofrio». Il presidente Marini insistette nel dire che sostanzialmente avrebbe dato la parola a colleghi di opposizione che formulavano proposte di modifica del calendario diverse da quelle già formulate dagli altri colleghi. Quindi

esempio guida di questa Presidenza del Senato. Per me il presidente Marini costituisce un faro di riferimento. L'ho detto fin dal primo momento di insediamento. Detto questo, presidente Zanda, dobbiamo trovare un punto d'intesa. Prego i Gruppi di opposizione di accettare questa proposta che consenta per le ore 14 - a meno che,

PdL).* Mi fa piacere vedere che adesso il presidente Marini gode di questa considerazione, ma mi dispiace dover ricordare che ciò non accadeva nella

Ricordo perfettamente le motivazioni della protesta che diedero luogo ad un famoso "lodo": cioè, si stabilì quali procedure adottare in occasione della discussione di provvedimenti

da un lato, per premiare un lavoro dettagliato ed un confronto serrato anche con le categorie professionali competenti

Quindi, lo assumo e lo propongo all'Aula e a lei, signor Presidente, come una priorità che ne confermerebbe il valore ed il significato e rafforzerebbe l'ordine naturale dei lavori delle Commissioni e dell'Aula. Non mi sembra che il provvedimento sulle intercettazioni contenga questi requisiti.

Presidente, la Commissione

legge predisposto dal Governo, insieme con altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, in materia anticorruzione. Non diamo affatto un giudizio particolarmente positivo sul disegno di legge di

che invece prevede norme molto più stringenti su una materia così delicata, cercando anche di recuperare un rapporto di fiducia con l'opinione pubblica che certamente negli ultimi mesi, dopo i gravissimi scandali che hanno colpito in particolare il settore della protezione civile, si è gravemente incrinato. Sarebbe un segnale molto positivo da parte delle istituzioni se il Parlamento

sarebbe di grande valore prevedere norme molto severe sulla incandidabilità - in particolare al Parlamento ma anche nei Consigli regionali, provinciali e comunali - di personalità che hanno commesso hanno commesso gravi reati e sono state condannate per vicende che suscitano grande allarme sociale. Sarebbe molto utile nei confronti dell'opinione pubblica anticipare questo disegno di legge anche in Aula e, nel contempo, rimandare l'esame

e l'*iter* parlamentare in Commissione sia completato assai rapidamente e si possa venire in Aula per affrontare questa delicata questione. [\*DELLA

insieme ad una mancata riforma organica della normativa sostanziale e processuale, impediscono di fatto di assicurarlo in tempi brevi e in modo efficace. La ragionevole durata del processo colpisce anche la ragionevole durata delle indagini preliminari. La discussione di una mozione sulla giustizia, in questi termini, consentirebbe di incastonare nell'ambito di una discussione politica

spesa per investimenti. Un allentamento del Patto di stabilità permetterebbe innanzitutto di mettere in moto opere medie e piccole, grazie alle quali verrebbe alimentata la piccola e media impresa italiana, in particolare nel settore dell'edilizia e del suo indotto. provocherebbe immediati benefici sul piano dell'occupazione, evitando il ricorso agli ammortizzatori sociali. Con quella mozione, una deroga mirata, regolata, monitorata al Patto, che consentirebbe la realizzazione e l'ultimazione di quegli interventi infrastrutturali

da un'elaborazione dei certificati di conto consuntivo del Ministero dell'interno di 104 Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, si evince che i residui passivi in conto capitale riferiti al 2007 ammontano a 1,5 miliardi di euro.

molti sindaci, di maggioranza e opposizione, hanno protestato e urlato che le loro amministrazioni sono ormai al collasso. Credo che calendarizzare questa mozione possa permettere finalmente

capita che lo Stato, a causa di un Patto di stabilità applicato in modo stupido, non paghi le forniture. In un Paese dove le spese per beni e servizi ammontano a circa 200 miliardi di euro, normalmente le imprese che erogano servizi e beni alla pubblica amministrazione aumentano i prezzi mediamente del 10-20 per cento in quanto, non incassando i soldi, aspettandoli per più di un anno, devono andare a scontare le fatture in banca. davvero vogliamo far diminuire la spesa pubblica dobbiamo iniziare a fare in modo che la pubblica amministrazione paghi in modo corretto ed entro 30-60 giorni, come avviene normalmente nel settore Solo questo potrebbe farci risparmiare, in termini di minore spesa pubblica, circa 20 miliardi l'anno. Questo è il modo per affrontare correttamente la crisi economica: il problema non si risolve trattando tutti allo stesso modo. In questo modo potremmo effettivamente

necessario che il Ministro della giustizia venga in Aula per spiegare al Paese quello che sta avvenendo realmente nel sistema giustizia italiano. Ci sono intere procure sguarnite di magistrati;

mentre sulle intercettazioni procediamo, e lo facciamo mettendo in serio pericolo tre delicatissimi versanti del sistema Paese: la sicurezza, signora Presidente, perché essa oggi è una vera priorità. L'avete cancellata, è uscita fuori dalla comunicazione, ma rimane. Oggi il sistema sicurezza, con la proposta che portate avanti sulle intercettazioni, non è più in grado di avanzare e ottenere risultati.

E così sulla libertà d'informazione: anche quella, una grande risorsa di un Paese avanzato, rischia di essere messa da parte. Ecco perché sulle intercettazioni non bisogna procedere, mentre si deve occupare l'Assemblea con provvedimenti e interventi in grado realmente di far crescere il nostro Paese e di renderlo più sicuro, più adatto alla lotta alle mafie e più libero nell'informazione.

entrare nel merito del provvedimento sulle intercettazioni in Aula senza aver prima compiuto un passaggio che ritengo di vitale importanza per il futuro del nostro Paese: penso che dobbiamo chiedere al ministro degli affari affari esteri Frattini di venire in Aula e riferire dei contatti che immagino abbia avuto in questi giorni, in queste ore, con l'Amministrazione americana, anche in considerazione della visita con il capo dello Stato Giorgio Napolitano sta effettuando a Washington, accompagnato, come Costituzione prevede,

Presidente, nel documento preparatorio della 46ª Settimana sociale dei cattolici italiani, un documento di grande rilievo e di grande interesse per il futuro del nostro Paese, si esprime preoccupazione rispetto al declino delle società occidentali e, in particolare, rispetto e, in particolare, rispetto al pericolo costituito da uno scenario nel quale la forza a disposizione di autorità che controllano società meno libere divenga superiore rispetto a quella di società più libere. È come se il tema della sicurezza e quello della libertà, che le società occidentali hanno saputo coniugare in maniera forte nel corso del Novecento, in questo momento tornassero ad essere elementi in contraddizione l'uno con l'altro. che il vice ministro della giustizia degli Stati Uniti, Lanny Breuer, nei giorni scorsi ha attirato l'attenzione del nostro Paese e della comunità internazionale. Ebbene, credo che su questo tema sia necessario ed opportuno un chiarimento rispetto all'opinione pubblica del nostro Paese ed alla comunità internazionale, che guarda con preoccupazione a questo passaggio. Per queste ragioni credo sia giusto chiedere al ministro Frattini di venire in Aula a riferire.

siamo di fronte ad un provvedimento che a nostro parere attenta ad un bene fondamentale per la comunità nazionale: la sicurezza pubblica. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno del giorno affinché prima del tema intercettazioni, su cui mi auguro vi sia un ripensamento del Governo e della maggioranza anche in rapporto alle proteste

una modifica costituzionale che attribuiva interamente queste materie alla competenza regionale. Come lei sa, quella modifica è stata poi respinta con il *referendum* del 2006; resta comunque ferma un'esigenza che noi, pur contrastando quella modifica, abbiamo sempre sostenuto, cioè che vi sia un raccordo molto forte tra istituzioni locali "Regioni" e sistema della sicurezza che faccia perno sulla polizia locale, che può avere un ruolo fondamentale in rapporto con gli altri apparati di sicurezza nazionale proprio per garantire, sul serio e senza propaganda, questo bene fondamentale per i cittadini. In Commissione affari costituzionali il provvedimento è già in uno stato molto avanzato: i colleghi Barbolini e Saia sono i relatori, volendo si potrebbe rapidamente concludere il suo esame per portarlo in Aula la prossima settimana. È quello che le propongo e le chiedo per fare una cosa buona per la sicurezza del Paese ed evitare, invece, che si compia un disastro.

alla possibilità, che ormai pare una certezza, che nella manovra finanziaria che sarà oggi ufficializzata dal Governo sia inserito un nuovo condono edilizio: quello che viene pudicamente chiamato «regolarizzazione delle case fantasma», ma che non sarebbe altro che il quarto condono edilizio generalizzato in 25 anni, dopo quelli del 1985 e i due varati da Governi Berlusconi nel 1994 e nel e nel 2003. Visto che, tra l'altro, da notizie che circolano non so quanto fondate, parrebbe che il primo ramo del Parlamento chiamato a discutere della manovra finanziaria sarà il Senato, io credo che sia assolutamente urgente che prima di iniziare questa discussione - di cui, ripeto, il nuovo condono edilizio è tema tra i più importanti - il Ministro dell'ambiente, nella giornata di lunedì o al più tardi di martedì, venga a riferire in Aula sull'impatto di questa misura dal punto di vista del rischio per centinaia di migliaia di italiani che vivono già oggi in aree a rischio sismico, vulcanico, idrogeologico e che aumenterebbero ulteriormente di numero se un nuovo condono edilizio, come è sempre avvenuto, innescasse una nuova ondata di abusivismo edilizio. In questa legislatura - lo faccio presente ai colleghi, a lei, signora Presidente, e al rappresentante del Governo - il ministro Prestigiacomo ha brillato per la sua assenza sistematica da quest'Aula: è stata assente anche quando si discuteva di provvedimenti che riguardavano in maniera diretta ed esclusiva le sue competenze ministeriali. Io credo che a questo punto sia non più rinviabile una sua presenza in Aula in Senato per dirci cosa pensa di questa misura inserita nella nuova manovra finanziaria e, in particolare, se ritiene che questa misura sia compatibile con la strombazzata in ogni occasione, del Governo e del suo Ministero di porre al centro delle proprie politiche e delle proprie scelte la messa in sicurezza del territorio. È di tutta evidenza, infatti, che un nuovo condono edilizio anziché contribuire alla messa in sicurezza del territorio contribuirebbe all'insicurezza del territorio e di tanti italiani.

di come morire, di come accettare o rifiutare delle cure nelle ultime fasi della nostra vita,

Quanto sarebbe persino più ecologicamente compatibile seguire ed adeguarsi a quelle che sono anche le nuove esigenze degli uomini e delle società, che cercano sempre più di

avevo presentato a metà del 2008 il disegno di legge n. per inserire nella nostra Costituzione la possibilità di un rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica. Avevo presentato questa proposta in seguito ad un rigonfiamento abnorme di una legge di conversione che aveva provocato le critiche del Presidente della Repubblica, il quale, all'atto della promulgazione, aveva segnalato il fatto che il testo fosse lievitato in maniera abnorme. Il Presidente della Repubblica ha posto di nuovo questo problema nella lettera con cui ha accompagnato la promulga della legge di conversione del decreto in materia

che colpisce l'Europa minandone le fondamenta e che rischia anche di declassare il nostro Paese; una crisi che per essere superata richiede una forte unità

allora, rivolgere una domanda al senatore Quagliariello, anche se ora non è in Aula: non crede che in questo sistema democratico, che per quanto imperfetto è il migliore che conosciamo, la dialettica, il dibattito e il confronto servano proprio, qualche volta, a cambiare idea o a trovare una sintesi che possa essere soddisfacente per tutti? tutti? Il Presidente della Repubblica richiama tutte le forze politiche ad una strategia solidale e responsabile: se non vogliamo che questi appelli se non vogliamo che questi appelli si perdano nel vento e se li vogliamo concretizzare, diamo spazio ad una dialettica che sia positiva e non negativa e di scontro, come purtroppo abbiamo visto anche in questi giorni.

di questa manovra tagli che non siano depressivi, ma che siano occasione di rilancio e di riqualificazione della struttura economica e sociale del nostro Paese, bisogna inserire all'ordine del giorno provvedimenti che cambino strutture

il calendario dei lavori del Senato non può che coincidere con il calendario dei problemi e delle attese del Paese. Che cosa è prioritario oggi per l'Italia? Ieri abbiamo approvato il provvedimento europeo per la Grecia. Bene. Ma il provvedimento sulle intercettazioni, che viene proposto nel calendario dell'Assemblea, peggiora le condizioni di sicurezza e di libertà dell'Italia. Guardo alla vita di milioni di italiani, di famiglie, di studenti. Guardo alla vita della scuola, che sta dentro la vita dell'Italia e che in questo momento è in profondissima sofferenza. Tra pochi giorni finisce un anno di scuola di grande difficoltà. A settembre ne comincia un altro: in quali condizioni organizzative noi non sappiamo. Non lo sanno le Regioni e gli enti locali che hanno potestà concorrente sulla materia, sull'istruzione. Abbiamo bisogno che ora, entro giugno - perché dopo non c'è più tempo - il ministro Gelmini venga qui e ci dica in cosa consistono effettivamente, sul piano organizzativo delle istituzioni scolastiche, delle classi e degli orari e dell'intero ordinamento, i tagli già previsti con la legge n. 133 del 2008. da quel momento non abbiamo più potuto discutere nulla con il Governo, con il Ministro. È come se avessero scippato insieme con questi soldi l'organizzazione complessiva di una delle strutture portanti della crescita e della vita del nostro Paese. Noi vogliamo che il Ministro venga a dirci come intende organizzare, nelle condizioni poste appunto da quella legge, la vita della scuola italiana per il prossimo anno e se non ci sia anche la necessità, se non la riconosca, di invertire la tendenza

dovere, il valore della scuola. Sono depositati da almeno un anno proposte di legge e due mozioni sulla materia che non sono mai state calendarizzate. Questo, a mio parere, è prioritario rispetto al resto. Il tempo per programmare il prossimo anno scolastico è questo per il Governo: è giugno, come tempo ultimo.

Presidente, chiedo di modificare il calendario dei lavori dell'Assemblea previsto per i prossimi giorni, seguendo le priorità che mi permetto di suggerire: nel senso di concludere l'*iter* di approvazione del disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense. Guardate, la maggioranza non lo vuole approvare questo provvedimento, altrimenti non lo porterebbe in quest'Aula a spizzichi e bocconi, dignità e una scarsissima attenzione nei confronti degli avvocati e del Paese, che attende questa riforma da molto tempo, per motivi a tutti noti. È inutile che ci prendiamo in giro:

Su questo tema la finanziaria del 2007 era intervenuta per disciplinare e meglio precisare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 2000, n. 38, con il quale era stato introdotto un nuovo sistema di indennizzo del danno permanente. Col disegno di legge, a mia prima firma, ma fatto proprio - ripeto - dal Partito Democratico, in primo luogo abbiamo ritenuto opportuno valutare come porre rimedio a quanto previsto nel decreto legislativo citato, ai sensi del quale, in caso di danno biologico, in luogo della rendita permanente prevista dall'articolo 66 del Testo unico, è invece previsto un indennizzo con un capitale *una tantum*, per le menomazioni di grado superiore al sesto ed inferiore al 16 Una tale previsione, Presidente, estromette molti degli invalidi del lavoro che non superano la soglia del 16 per cento da una serie di servizi che spettano ai titolari di rendita permanente, facendo venire meno l'impiego dell'INAIL alla presa in carico globale dell'infortunato sul lavoro. Al fine di evitare questa situazione, il disegno di legge dispone che godano dell'erogazione delle rendite gli invalidi con grado di inabilità superiore all'11 per cento. In secondo luogo, signora Presidente, questo disegno di legge provvede ad attribuire una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi che siano atti atti a ridefinire la disciplina dell'indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Fra i vincoli posti al Governo nell'esercizio della delega vi sono quello di prevedere una modifica sulla base di calcolo delle quote integrative spettanti all'infortunato per il coniuge e i figli a carico, tenendo conto dell'intero importo delle quote di rendita, e quello dell'applicazione del criterio della media giornaliera nel settore industria

così male nato come quello sulle intercettazioni telefoniche, che tante divisioni sta creando nel nostro Paese. Ne cito uno. È terminato in Commissione l'*iter* del disegno di legge di riforma sull'università, l'Atto

infatti, l'Italia deve ripartire, riparte accumulando conoscenza, riparte riqualificando gli studi, riparte investendo nell'università. Invece, noi arriveremo all'inizio del prossimo anno accademico senza una legge e con il cappio al collo di un ulteriore taglio di risorse per l'università che si commisura in 1.300 milioni. Questa è

calendarizzato al più presto. È uno dei modi per uscire dalla pesantissima crisi nella quale ci troviamo.

come tutti sanno, sta attraversando una grave crisi economica e finanziaria, con effetti pesantissimi sulle imprese e sull'occupazione. Nel primo quadrimestre di quest'anno abbiamo registrato circa 3.000 fallimenti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno passato; dall'inizio della crisi, nell'ottobre 2008, abbiamo perso circa 700.000 posti di lavoro e nello stesso periodo sono stati collocati in cassa integrazione più di un milione di lavoratori e lavoratrici. Dopo avere lungamente negato la gravità della crisi, l'altro ieri il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, ha dichiarato che «ci aspettano» - cito testualmente - «sacrifici pesanti, sacrifici molto duri, sperando che questi sacrifici siano provvisori». Ieri il Consiglio dei ministri ha varato una manovra economica rilevante, una manovra che prevede tagli indiscriminati e senza nessuna equità, una manovra dal carattere economico recessivo. Le riforme, a partire da quelle sociali, vengono ancora rinviate

e persino, ultimo emendamento del Governo, il ripristino del licenziamento in forma orale: davvero un salto all'indietro che non si era davvero mai visto. si attaccano questi diritti, domani, come ha annunciato la settimana scorsa in questa Aula il ministro Sacconi, il Governo si appresta a svuotare lo Statuto dei diritti dei lavoratori. Signori del Governo, Signori del Governo, se davvero volete aprire un confronto con le opposizioni, come ha giustamente auspicato nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, dovete sgombrare il terreno

sul lavoro. In quella discussione il Governo si impegnò a dare una risposta a queste tragedie continue, a queste cosiddette morti bianche. In particolare, in merito ad un aspetto,

fare valutazioni sulle tragedie che viviamo e continuare il solito andazzo per far fronte alle procedure che interessano a Berlusconi e alla sua

in quest'Aula. Io mi permetto di segnalarle uno. Chiedo che, ai sensi dell'articolo 105 del Regolamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Abbiamo i petrolchimici di Porto Marghera, di Brindisi, di Taranto, di Priolo e di Gela. Abbiamo aree urbane industriali, come Napoli orientale, Trieste, Piombino, La Spezia, Brescia, Mantova. Ci sono vere e proprie emergenze sanitarie nel Paese. Non sappiamo come avverrà la gestione dei materiali provenienti dalle attività di bonifica. Non sappiamo quanto la malavita organizzata si fionderà su questa attività. Non sappiamo i costi delle bonifiche. Non sappiamo quali siano i contenziosi amministrativi tra gli gli enti di controllo, che sono tanti e impediscono la bonifica di tali aree. Non sappiamo come avverrà la gestione dei sedimenti contaminati. Non sappiamo dove siano finiti gli smaltimenti illegali. E ce ne sono molti. Non sappiamo a che punto siano i disastri ambientali conseguenti. Il ministro Gelmini è favorevole ad allungare le vacanze, vacanze, ma io mi chiedo: gli studenti di Crotone, come faranno ad andare al mare con l'area contaminata di Pertusola Sud - un'area un'area contaminata da oltre 70 anni - che non sappiamo quali effetti abbia sul bel mare della Calabria? Non sappiamo quanti inquinamenti ci siano a seguito di incidenti dolosi. Pensiamo a quel che è avvenuto per l'inquinamento del Lambro. Pensiamo ai nuovi danni derivanti dalla omessa bonifica. Ancora, non sappiamo quale sia il livello di contaminazione dei suoli e delle acque conseguente soprattutto alle attività dei petrolchimici. A questo punto credo che sia tempo che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare venga a riferire in quest'Aula e chiedo che il Senato possa votare una risoluzione su tale argomento, che riguarda la salute e la sicurezza dei cittadini di oggi e di domani, senza contare i gravi danni già avvenuti in tutte queste aree a carico dei lavoratori e delle loro famiglie.

Tra queste, c'è il disegno di legge n. 784 («Misure urgenti a sostegno della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale nonché deleghe al Governo in materia di tutela della maternità delle lavoratrici

Abbiamo già svolto numerose, interessanti audizioni e tutti i soggetti auditi ci hanno chiesto di procedere in maniera spedita. In questo momento di crisi che ha inferto una ferita profonda, soprattutto sui livelli occupazionali, il tema del lavoro femminile certamente è una priorità, e non riguarda soltanto le donne o l'economia, ma la società nel suo complesso. È infatti inerente anche ai temi dei diritti e dei servizi sociali, all'organizzazione familiare, al grave calo demografico del nostro Paese. Siamo convinti che il sostegno alla partecipazione al lavoro delle donne presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese nonché strumento essenziale per la crescita e la competitività del nostro sistema produttivo. produttivo. Cerchiamo di dare dei segni tangibili all'esterno che dimostrino che ci stiamo occupando dei bisogni e dei problemi del Paese. In questo modo forse riusciremo anche a dare un contributo per colmare il *gap* esistente tra le istituzioni e i cittadini, e forse anche a dare una risposta alla campagna di discredito delle istituzioni, e del Parlamento in primo luogo, di cui oggi siamo in qualche modo vittime.

Signora Presidente, anch'io chiedo di modificare l'ordine dei lavori dell'Aula della prossima settimana per inserirvi gli adempimenti al Regolamento per l'implementazione del Trattato di Lisbona che, tra l'altro, competono alla Presidenza di questo Senato. Si tratta di adeguamenti necessari per arricchire gli strumenti di intervento del Senato nelle decisioni comunitarie. Sono passati ormai sei mesi dall'entrata in vigore del Trattato e circa quattro mesi dalla conclusione dei lavori del Gruppo appositamente predisposto dalla Presidenza. Arrivare al più presto a questi primi adeguamenti regolamentari è necessario per assicurare l'autonomia istituzionale ed organizzativa del Senato nel processo di integrazione istituzionale e politica dell'Unione, ieri da più parti invocata nel dibattito sulla Grecia. Vede, Presidente, noi insistiamo su questo perché riteniamo che oggi per il nostro Paese la priorità non sono le intercettazioni, ma è l'Europa e la drammatica crisi degli Stati nazionali. Per questo insistiamo. Infatti, oggi, la prima cosa che spicca agli occhi di tutti, in Italia e in Europa, e che preoccupa anche molto, è che l'Italia è l'unico Paese europeo dove non si discute di Europa, della sua crisi e del suo futuro. Per mesi avete sottovalutato la crisi economica. Adesso che vi siete svegliati le misure mirano a giocare la sola carta degli interventi sui conti pubblici, sicuramente necessari, ma che non costituiscono i presupposti per il futuro. Anche per questo chiediamo l'iscrizione all'ordine dei lavori dell'Aula dell'adeguamento del Regolamento sul Trattato di Lisbona. Si tratta di un passo urgente da compiere perché utile per il sistema Italia e per contribuire alla costruzione di uno spazio politico europeo. Grazie Presidente, come vede ho mantenuto il

dalla discussione e dall'approvazione, nelle forme in cui è stato esaminato in Commissione, del disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche. Mi preme sottolineare il fatto che le mie preoccupazioni attengono soprattutto ai rischi per la sicurezza dei cittadini e i rischi per la legalità dei mercati. Si configura una situazione in cui sarà possibile una maggiore libertà nel compiere gravi reati societari; i reati contro il patrimonio e i reati fiscali non saranno intercettabili e non saranno intercettabili e quindi saranno assai più difficilmente contrastabili e da ciò deriverà un detrimento pesante per la sicurezza delle nostre imprese e per la libera competitività fra di esse. In questo

tutte le proprie energie e tutto il proprio tempo, mettendo all'esame dell'Aula proposte legislative che, anche con diversa portata, possano contribuire a creare i presupposti per portare il nostro Paese fuori dalla crisi in un'ottica di sviluppo e non di mera sopravvivenza. Questa è la ragione per la quale chiedo la calendarizzazione urgente del disegno di legge n. 1864 in materia di pari opportunità, che ho sottoscritto insieme alla senatrice Vittoria Franco e che dispone misure in parte analoghe a quelle previste dal disegno di legge n. 1719 a prima firma della senatrice Germontani del Gruppo Questi disegni di legge muovono dal presupposto che il sostegno alla partecipazione al lavoro delle donne sia un fattore determinante, come veniva detto, per la crescita economica e civile, nonché per l'equilibrio democratico del nostro Paese. È noto che i dati relativi alla presenza delle donne nella *governance* delle imprese del nostro Paese sono drammatici: l'Italia è al 29° posto su 33 Paesi censiti per numero di donne presenti nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa. cento degli amministratori sono donne, contro l'11 per cento della media europea; dopo di noi vengono solo Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo, Paesi che certo non si trovano in condizioni ottimali in questa fase di crisi. E poiché è dimostrata la sussistenza di un nesso strettissimo tra la parità lavorativa e la partecipazione delle donne ai processi decisionali, chiedo di calendarizzare questi disegni di legge, che peraltro...

proprio ieri in Commissione sanità sono stati esaminati e illustrati tutti gli emendamenti a un testo condiviso da maggioranza e opposizione, un testo che riguarda le malattie

due milioni le persone che soffrono di queste malattie, ed il 50 per cento sono bambini, bambini che soffrono fin dalla nascita. Ed allora mi chiedo: questo Parlamento si deve occupare delle intercettazioni o si deve occupare di questi bambini, delle loro famiglie, delle difficoltà che affrontano? Sono ben quattro legislature che al Senato della Repubblica si discute di questi problemi

partiti sono sempre più ricchi in un Paese sempre più povero, si dice. Abbiamo il diritto e il dovere di proporre controriforme, proposte nuove e serie

È una legge relativamente giovane, si dirà; sono forse troppo pochi 68 anni per adeguare una normativa ai grandi cambiamenti del settore: potremmo aspettare anche il 70° anniversario,

Potrebbe essere utile a milioni di cittadini che hanno visto la disciplina rimanere immutata e le condizioni, le fattispecie, la realtà di ogni giorno cambiare invece...

sono talmente tante le proposte che stiamo avanzando che basterebbe che quest'Aula ne accogliesse qualcuna. Per affetto, per amore - che credo condiviso in questa Aula e fuori di qui - ricordo che che questa mattina risultano essere tante le iniziative, anche parlamentari, utili al Governo che non vengono mai prese in considerazione. Mi riferisco alla proposta

Vuol dire che davvero né allora, né ora si riconosce la dignità, l'importanza della Croce Rossa Italiana anche nel contesto internazionale. Eppure è una delle più efficaci ed effettivamente inserita nel contesto internazionale. Questo Governo, se davvero vuole esprimere

può fare, questa che state facendo voi della maggioranza è sicuramente di una curiosità e di una fantasia straordinarie. Avevate depositato questo provvedimento da un sacco di tempo, avete deciso di riesumarlo forse nel momento politicamente meno adeguato e adatto, adesso cercate di forzarlo, probabilmente verso un voto di fiducia già la settimana prossima. Questo pare francamente esagerato rispetto alle urgenze che ha il Paese. Tanto più che quelli che ponete non sono argomenti che non abbiamo contemplato: quello dell'equilibrio tra il diritto del cittadino a non essere

eccessi, che va ritrovato un nuovo equilibrio, che le intercettazioni non possono essere una scorciatoia per azioni giudiziarie che costruiscono castelli accusatori che cadono al primo giudizio, così come sappiamo che il giornalismo non può semplicemente essere il *report* di una intercettazione, ma deve approfondire. Esiste un disegno di legge, tra l'altro già approvato dalla Camera, proposto dal Governo Prodi la scorsa legislatura: c'è spazio per un dialogo, per trovare in questo momento un testo condiviso,

un provvedimento - tra i tanti che sono stati citati, ne cito un altro che mi sta a cuore - quale la riforma degli ordini professionali non medici? Si tratta di un provvedimento che è pronto per essere approvato; in Commissione sanità potremmo lavorare molto velocemente perché

Presidente, colleghi, in questi giorni la preoccupazione è molto grande in merito alla crisi economica. Ci si chiede come possa fronteggiarla il nostro Paese, quale sia il suo capitale per farlo: il capitale che può mettere a disposizione è la credibilità.

La stessa competitività sui mercati internazionali non la si ottiene, nell'epoca dell'economia della conoscenza, investendo sull'istruzione e sull'aiuto alle famiglie perché i propri figli possano crescere ed essere educati ed istruiti al pari dei grandi Paesi europei? Il nostro è il Paese che ha il tasso demografico più basso al mondo (la CEI parla di suicidio demografico), ha il tasso di povertà minorile più elevato in Europa, ha il tasso di dispersione scolastica più elevato e anche nei dati OCSE-PISA riceve i livelli più bassi. Mentre la Gelmini parla - ed è veramente incomprensibile come un Ministro responsabile possa farlo,

dalla presidente Finocchiaro circa la necessità di far slittare un provvedimento sbagliato e certamente da rivedere, quello sulle intercettazioni, avendo noi alcune

esemplificata da quello che ha dichiarato recentemente il presidente Obama in merito alla alla necessità per un Paese evoluto di investire in tecnologie, banda larga, ricerca. Lo slogan «banda larga per tutti» non è solo una chimera, ma è oggi un'assoluta un'assoluta e indispensabile questione per le società postfordiste dell'economia della rete. Solo così anche la crisi economica tanto grave può trovare forme di risposta non congiunturali o effimere; solo così si può investire sul futuro e sui giovani che, proprio attraverso la tecnica digitale, oggi hanno un'altra possibilità di immergersi nella conoscenza.

lontanissimi dal 3 per cento di Lisbona. Dunque, cosa si attende a discutere come in tutti i Paesi evoluti della rete, della nuova forma della comunicazione e della conoscenza? L'Italia oggi è un Paese che rischia di essere arretrato e di essere messo fuori dal consesso più evoluto. Tra l'altro, proprio il disegno di legge Alfano sulle intercettazioni mette un altro cappio alla rete - ed è un motivo in più per rinviarne la discussione

per le ragioni che qui sono state illustrate dalla senatrice Finocchiaro innanzi tutto, ovverosia la necessità di discutere in quest'Aula di un testo che sia nelle nostre mani, quindi per il rispetto che tutti noi

Ecco allora che vorrei ricordare una iniziativa parlamentare di cui sono la prima firmataria (ma ce ne sono anche altre su questo argomento, che giacciono in Parlamento) a proposito di un tema di cui non si discute da molti anni e che, invece, è di estrema attualità. Chiedo che venga iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2162

c'è e quanta parte del corpo elettorale sono le donne. L'ultima volta che il Parlamento ha discusso di questo tema è stato nel 1985, con le vituperate quote rosa, di cui tanto si parlò per poi non farne nulla. farne nulla. L'unica Regione che ha portato un risultato diverso è stata la Campania che, con una nuova legge elettorale, ha visto l'elezione di 15 donne, senza quota, con la sola possibilità di

personalmente che l'attività di un parlamentare debba alimentarsi costantemente del contatto con i territori e le comunità. Molto spesso ciascuno di noi, anche in ambiti geografici differenti da quello di cui è espressione, si trova ad essere investito di questioni e di problematiche che riflettono altrettante legittime

a condizione che - ragionevolmente aggiungo io - se ne faccia un uso discreto e misurato. 1050 a risposta scritta. Le risposte orali da parte del Governo sono pervenute solo in minima parte; le risposte complessive del Governo ad interrogazioni scritte ed orali presentate dal gruppo del Partito Democratico al Senato dall'inizio della legislatura sono 619. Vorrei ricordare che l'articolo 148 del Regolamento del Senato prescrive che le interrogazioni a risposta orale siano poste all'ordine del giorno non oltre il quindicesimo giorno dalla loro presentazione. Anche con riguardo alle interrogazioni a risposta orale in Commissione, disciplinate dall'articolo 147 del Regolamento, a non mi pare che vi sia un particolare attivismo da parte del Governo, come abbiamo avuto più volte occasione di rilevare in Commissione agricoltura. È evidente che il rinvio *sine die* delle risposte su problemi specifici vulneri e addirittura vanifichi la natura e le funzioni stesse delle interrogazioni e delle interpellanze. In altri termini, vi è una giacenza molto rilevante di interrogazioni inevase. Se non recuperiamo un rapporto più corretto di interlocuzione tra l'Assemblea legislativa ed il Governo non renderemo renderemo un buon servizio all'istituzione parlamentare, perché la allontaneremo sempre più dai cittadini. Noi parlamentari abbiamo il dovere di evitare che ciò accada che ciò accada o che si materializzi un disegno, che da troppo tempo ha preso corpo e forma, di sostanziale, progressiva, lenta e graduale,

perciò, la modifica del calendario dei lavori, avanzando la richiesta di due giorni di seduta che il Senato dovrà dedicare con assoluta tempestività al sindacato ispettivo. Signora Presidente, le notizie di questi giorni, e non solo di questi ultimi giorni, ci dicono che la casa brucia. È in crisi l'economia, è in crisi il settore industriale, è in crisi il mercato del lavoro, ma in quest'Aula sembra che la priorità non sia spegnere l'incendio, ma occuparsi d'altro. Un esempio: mai come oggi, nel pieno della crisi, la carenza infrastrutturale del nostro Paese viene denunciata come principale causa dello stato malandato della nostra economia. Ebbene, da diversi mesi in 8a Commissione stiamo discutendo una legge fondamentale per il miglioramento delle infrastrutture del nostro Paese. Parlo del disegno di legge che, unificando e coordinando i testi dei disegni di legge nn. 143, 263 e 754, determina i nuovi principi in materia di porti e i nuovi criteri per ripartire compiti e funzioni tra autorità marittime e autorità portuali. Chiedo che tale disegno di legge sia calendarizzato al più presto in quest'Aula, essendo esso molto più urgente e necessario di una legge sulle intercettazioni ingiusta, mal congeniata e lesiva delle libertà individuali. Le infrastrutture e, in un Paese come il nostro, i porti in primo luogo sono fondamentali per determinare la capacità competitiva del sistema produttivo. Oggi l'Italia, nonostante per vocazione naturale sia un Paese che guarda al mare come fonte di ricchezza, è dal punto di vista dell'efficienza del suo sistema portuale agli ultimi posti in Europa. Per questo motivo, riteniamo più utile che quest'Aula si occupi nei prossimi giorni di questo provvedimento piuttosto che di quello sulle intercettazioni. la mia proposta è di aggiornare l'iscrizione del provvedimento di cui stiamo trattando alla prima seduta successiva alla pausa estiva, e motiverò rapidamente il perché di questa richiesta. Veda, Presidente, se Demostene fosse vissuto ai giorni nostri anziché ai tempi di Filippo avrebbe trasformato il suo severo monito «*oportet ut scandala eveniant*» nel più attuale «*oportet ut scandala inveniant*».

siano improntate all'obiettivo di intralciare il corso della giustizia e di impedire l'accertamento della verità. Sostanzialmente, con il pretesto della tutela della *privacy* e dei diritti dei cittadini, si intende effettivamente porre ostacoli all'accertamento della verità.

attraverso l'introduzione nell'ordinamento di norme che, ad esempio, individuino e consentano la tracciabilità degli atti soggetti a segreto istruttorio, così da individuare adeguatamente i responsabili di eventuali violazioni del segreto istruttorio stesso. Questo è l'obiettivo che abbiamo perseguito con un lavoro intenso, compiuto in Commissione per circa un anno, Presidente. Sicché, nel momento in cui si discute di tagli agli sprechi, noi riteniamo che sia fondamentale cercare di tagliare lo spreco più odioso per un'Aula parlamentare: lo spreco del lavoro istituzionale. Questa maggioranza si propone di calendarizzare un provvedimento che - ripeto - ha impegnato la Commissione giustizia, autorevolmente presieduta dal collega Berselli, per circa un anno nel breve volgere di soli due giorni, così impedendo a questo Parlamento di corrispondere ai propri doveri fondamentali e di avere soprattutto rispetto per se stesso, per questo organo costituzionale rispetto per i cittadini e per il Presidente della Repubblica, che, così come ci ricordava il collega Ceccanti, ancora una volta ha sollecitato la maggioranza ed il Governo*...

da anteporre a questo dibattito sulle intercettazioni telefoniche, dibattito che consideriamo, appunto, non così urgente e rispetto al quale opponiamo un nostro giudizio di contrarietà nei termini di una corretta opposizione, senza atteggiamenti particolarmente ostili alla procedura parlamentare. Ma dentro la stessa, vogliamo vogliamo esprimere il nostro dissenso in termini positivi e propositivi, cercando ed invocando la collaborazione anche della maggioranza per una diversa composizione dell'ordine del giorno. Mi associo a quanto ha chiesto il collega Ranucci, appoggiandomi ad un'altra delle mozioni presentate già il 22 luglio 2009, la mozione n. 241, che prendeva lo spunto dalla questione, ormai a tutti noi nota, del cosiddetto Patto di stabilità, che trasforma in molti casi i nostri enti locali in sistemi incapaci di poter produrre una amministrazione adeguata ai bisogni dei nostri cittadini. Il problema è urgente perché, rispetto alla manovra che si annuncia, sappiamo già dalle anticipazioni di stampa che sono programmati altri tagli agli enti locali, che è programmato un altro livello di restrizione per il Patto di stabilità, e mentre sappiamo questo, sappiamo anche che in sedi parallele, nel quadro delle attività parlamentari, stiamo avvicinandoci ad una discussione che rischia davvero di essere paradossale, quella sul cosiddetto federalismo fiscale, che dovrebbe trasmettere alla pubblica opinione l'idea di un quadro molto diverso dalla realtà, in base al quale gli enti locali avrebbero chissà quali possibilità di intervento e di manovra. Ora, è evidente che, se rispetto all'urgenza vera, che è quella di affrontare la crisi economica e finanziaria con un disegno chiaro, non agiamo in anticipo, facendo chiarezza su quello che stiamo facendo qui in Parlamento, una volta parlando separatamente ed in modo segmentato di una questione, cioè il federalismo fiscale,

Signora Presidente, come già richiesto da molti altri colleghi, anch'io chiedo una modifica dei lavori dell'Assemblea e di calendarizzare prioritariamente provvedimenti che rispondano maggiormente alle esigenze del Paese nell'attuale fase di crisi economica e sociale, una crisi che rischia di rompere anche il già fragile tessuto di solidarietà che lo tiene ancora unito. Alla Commissione attività produttive è stato assegnato qualche mese fa il disegno di legge che intende promuovere misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, attraverso buone prassi gestionali, produttive e comportamentali che favoriscano una maggiore tutela dell'ambiente, uno sviluppo durevole, la salvaguardia delle comunità nelle quali è inserita l'impresa, la crescita professionale degli occupati lungo tutto l'arco della vita, la buona organizzazione del lavoro, con ricadute benefiche sulla gestione della famiglia e dei figli, l'eguaglianza delle opportunità, l'inserimento sociale e il rispetto degli utenti e dei consumatori. Una gestione responsabile e consapevole delle trasformazioni non può che avere effetti positivi a livello macroeconomico. Al di là del perimetro interno, la responsabilità sociale dell'impresa coinvolge oltre ai lavoratori dipendenti e agli azionisti, i *partner* commerciali, i fornitori, i clienti, i poteri pubblici e le organizzazioni non governative che rappresentano la comunità locale e l'ambiente. In Italia finora il tema della responsabilità sociale delle imprese, almeno nella legislatura in corso, non è stato al centro del dibattito politico. A questo argomento sono stati dedicati apprezzabili approfondimenti, ma finora non si riscontrano significativi interventi per affrontare il dibattito della diffusione delle buone prassi comportamentali nell'ambito del nostro sistema imprenditoriale. Per questo ritengo opportuno che questo disegno di legge venga discusso, in sostituzione del provvedimento sulle intercettazioni del quale, francamente, non si avverte davvero l'urgenza.

per suggerire a quest'Aula di lavorare e di confrontarci su temi - come diceva prima la capogruppo Finocchiaro - di cui sicuramente il Paese ha più bisogno rispetto al provvedimento sulle intercettazioni. Nel mio caso, propongo di calendarizzare il disegno di

anche quella fatta propria dalla nostra Costituzione. Il valore persona umana costituisce la parte caratterizzante l'ordinamento giuridico, tanto da garantirne l'armonia e l'unitarietà di intenti e la famiglia, nel suo aspetto sociale e nel suo riflesso giuridico, si lega inscindibilmente inscindibilmente all'esistenza, alla dignità e alla personalità di ciascuno dei suoi componenti. Da tempo nei vari Paesi europei la tendenza è a una completa equiparazione tra tutti i figli, senza ulteriori qualificazioni. Le convenzioni europee che si sono succedute sui diritti dell'uomo e del fanciullo, raccomandazioni comunitarie ed altro, disegnano un unico quadro rispetto al quale l'Italia è ancora arretrata. La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo tratteggia la famiglia come un organismo che presuppone lo sviluppo della personalità dei suoi componenti sulla base dei principi di pari dignità, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà. Da qui discendono alcuni principi, tra i quali si possono sicuramente menzionare quelli relativi alla tutela dei figli, per se stessi, cioè in quanto individui nati, e alla pari dignità dei figli naturali rispetto ai figli legittimi. In Italia, e malgrado il principio di uguaglianza sancito nel 1975 dalla riforma del diritto di famiglia, c'è ancora una differenza tra i diritti dei figli legittimi e quelli dei figli cosiddetti naturali, meglio dire nati fuori dal matrimonio, bambini che non hanno diritto ad una piena e legittima parentela, a un nonno, a uno zio, nella loro funzione pienamente legale. Si può pensare ciò che si vuole delle scelte individuali di formare o meno una famiglia fondata sul matrimonio, e sono tutte opinioni rispettabili, ma non si può che il principio che i minori, i bambini abbiano diritto ad una pienezza della parità del riconoscimento umano, affettivo e giuridico.

pur trattandosi di un tema molto grave, urgente ed anche molto dibattuto su una certa letteratura pubblicistica che sta diventando anche molto importante: come i *media* rappresentano le donne,

che equivale all'immagine del corpo femminile muto, compiacente verso i desideri maschili, e della donna dedita pressoché esclusivamente a curare la sua bellezza ed il suo corpo. Nessuna visibilità a donne che invece hanno successo nella ricerca scientifica, nell'imprenditoria, nella medicina e nella cultura e, vorrei aggiungere, anche nella politica. La vicenda che ha visto due giornaliste RAI come Tiziana Ferrario e Maria Luisa Busi di fatto estromesse dalla conduzione del TG1 dimostra che

l'impegno di un esplicito e chiaro contrasto alle discriminazioni ed agli stereotipi di genere, a favore del rispetto della dignità delle donne, che è un bene di civiltà e di democrazia. Nella nostra mozione noi sia impegnato a promuovere campagne di informazione finalizzate alla diffusione ed alla valorizzazione del lavoro e delle opere delle donne nei campi dell'arte, della cultura, della scienza e della politica e ad adottare campagne di sensibilizzazione nelle scuole, in particolare nella scuola secondaria, per aiutare i giovani a difendersi dai messaggi discriminatori nei confronti delle donne e per evitare così il perpetuarsi di stereotipi che danneggiano le donne e il ruolo femminile nella società. *(Applausi Signor Presidente, credo che in una giornata come questa non vi sia nessuna Aula parlamentare in Europa che non si stia occupando della crisi economica, dei mercati finanziari, della crisi che si riverbera sul sistema delle imprese, dei disoccupati che nascono e delle imprese che stanno chiudendo. Credo che in nessun Parlamento europeo si possa consentire, in giornate come queste, di non affrontare temi nodali, quali, ad esempio, quello dell'accesso al credito per le piccole e piccolissime imprese, che si dimostra nel nostro Paese più ancora che in altri il vero aspetto di problematicità in una fase di crisi che unisce gli aspetti economici e produttivi a quelli della chiusura del credito e della totale dipendenza delle imprese, soprattutto le piccole e piccolissime, dalle banche.

Grazie si ritorni a dare priorità totale all'emergenza economica del Paese ed in questo senso si calendarizzi un disegno di legge inerente allo sviluppo di strumenti finanziari di mercato per il sostegno delle piccole imprese, in particolare di quelle in difficoltà e in crisi. Perché strumenti finanziari di mercato? Perché la piccola impresa italiana è costretta al 90 per cento a fare ricorso esclusivamente al fido di conto corrente, cioè alla forma più esposta, più gravosa e costosa di accesso al credito. Strumenti più innovativi che possono mobilitare il risparmio territoriale, delle famiglie, la nascita di fondi chiusi, che possono contemporaneamente veicolare risorse di natura finanziaria e manageriale verso le piccole imprese e le loro reti (esempi ve ne sono di questa possibilità), dovrebbero essere facilitati e messi nella condizione di divenire competitivi i nostri sistemi economici. in giornate come queste sarebbe ora di raccogliere le idee su come rilanciare la nostra economia in modo innovativo e non assistito. Facciamo tutt'altro; è un peccato per questo mondo straordinario di imprese, è un peccato per un mondo straordinario dell'economia italiana. Peccato, stiamo facendo dell'altro.

anch'io chiedo di cambiare il programma dei lavori e di togliere dal calendario di lunedì il disegno di legge sulle intercettazioni, la cui pericolosità è stata ampiamente segnalata in quest'Aula. È un disegno di legge che limita ingiustificatamente lo strumento delle intercettazioni, allunga i tempi delle indagini con inutili formalità, formalità, porta ad una non tutela della *privacy*, impedisce ai cittadini di essere informati sul malaffare durante tutto il corso delle indagini, quindi per anni. Credo onestamente che sia difficile contestare quel che molti colleghi hanno detto, cioè che la priorità di oggi del nostro confronto dovrebbe essere la gravissima situazione economica del Paese, che in quest'Aula sarebbe assolutamente necessaria una discussione politica assai seria e approfondita sulla situazione reale della nostra economia, quella stessa discussione che finora è mancata poiché la maggioranza e il Governo hanno prima pervicacemente negato l'esistenza stessa della crisi, poi l'hanno minimizzata, poi hanno sparso a piene mani ottimismo circa il fatto che l'Italia vivesse comunque una condizione di favore rispetto all'universo mondo, infine hanno detto che eravamo già fuori dal tunnel. Un atteggiamento irresponsabile che viene spazzato via dalle stesse parole del sottosegretario Letta dell'altro ieri. C'è bisogno di discutere di questo. Ci sarebbe bisogno di discutere di questo, della situazione reale della nostra economia, del nostro assetto produttivo, dell'occupazione, dei redditi, di chi lavora, dei precari, dei giovani che si interrogano angosciati sul proprio futuro. Di questo c'è bisogno. Questo si attende da noi il Paese. Di questo vuol sentirci parlare proprio quando sui cittadini si sta abbattendo una dura manovra economica. Per questo io chiedo che si possa discutere il disegno di legge n. 1110, che immette in una fase di crisi come questa gli elementi di riforma necessari.

*(PD)*. Signora Presidente, anch'io chiedo di modificare il calendario dei lavori dell'Aula seguendo una diversa priorità rispetto a quella proposta. È per questo che chiedo di inserire al posto del disegno di legge sulle intercettazioni l'insieme dei disegni di legge n. 1079 e altri in materia di prostituzione;

strombazzato all'esterno come risolutore di tanti gravi mali che affliggevano l'Italia. Si diceva: «Il presente schema di disegno di legge è stato predisposto per contrastare efficacemente il fenomeno della prostituzione ed il suo sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali». Nello specifico voleva affrontare la prostituzione di strada, facendo riferimento a misure che in primo luogo tutelino la dignità, i valori della persona umana e la sua libertà di determinazione ed in secondo luogo prevengano le cause di un diffuso allarme per l'ordine pubblico e la sicurezza. gli stessi contenuti che ci vengono presentati per motivare l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge sulle intercettazioni. In più, si diceva che con l'introduzione del reato di prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico si mirava ad eliminare la prostituzione di strada come fenomeno di maggior allarme sociale e contemporaneamente si voleva contrastare lo sfruttamento della stessa in quanto è soprattutto in luogo pubblico che si perpetrano le più gravi fattispecie criminose finalizzate allo sfruttamento sessuale. Si parlava poi della prostituzione minorile e si cercava di risolvere i problemi che le ordinanze di sicurezza dei sindaci avevano introdotto. Ma segnalo soprattutto che i lavori erano terminati:

Infine, non vorrei mai, e parlo per assurdo, che i cittadini pensassero che questa omissione della calendarizzazione del provvedimento sulla prostituzione fosse frutto di resipiscenza, proprio così, di una qualche resipiscenza di qualche utilizzatore finale pentito.

Le elezioni politiche sono state vinte anche speculando sulla sicurezza, cavalcando, mi si consenta, in modo squallido, alcune violenze carnali - penso alla povera signora Reggiani - e seminando di conseguenza terrore. Questo ha pagato, ma ovviamente nulla è cambiato. Quante violenze, quanti altri gravi reati sono avvenuti? Non è aumentata, sia ben chiaro, la sicurezza, ma è diminuito lo spazio che certa stampa asservita dedica al problema. Allora si è messo mano a leggi demagogiche quanto vane. Mi chiedo che fine hanno fatto le ronde e le strutture carcerarie. Le case circondariali oggi contengono 65.000 detenuti a fronte dei 45.000 che potrebbero contenere. Dove entreranno i cosiddetti clandestini, per i quali la demagogica norma prevede l'arresto ed il processo per direttissima? Parole e ancora parole.

stati pubblicizzati arresti di mafia che, sia ben chiaro, sono sempre avvenuti con qualunque Governo, di destra e di sinistra. sono ancora tagli. Questi sono gli argomenti prioritari, e non la limitazione delle intercettazioni che, oltre ai fondi, taglia anche gli strumenti di indagine che, mi sia consentito di affermare, sono di fondamentale rilevanza. Chiedo quindi che il Ministro dell'interno venga in Aula per chiarire come intenda gestire questa nuova drammatica situazione e limitazione di fondi, prima ancora di calendarizzare il provvedimento sulle intercettazioni. Spero che il ministro Maroni, sempre attento ai suggerimenti dell'opposizione, voglia cogliere questa richiesta che potrebbe tranquillizzare gli operatori di polizia e la gente comune, delusa delle tante promesse non rispettate.

il disegno di legge n. 1813 recante disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva. prima di tutto da me, ma è stato sottoscritto anche da numerosi altri colleghi; vorrei ricordare, tra gli altri, il collega Barelli del PdL, il collega Giambrone dell'Italia dei Valori, il collega Pittoni della Lega Nord, il collega D'Alia dell'UDC,

pubblica e da tutti i colleghi che si occupano di sport, che è stato preceduto da un'indagine conoscitiva che ha riconosciuto il grande valore sociale dello sport dilettantistico, con 95.000 società sportive che rischiano di pagare l'impatto della crisi economica con il venire meno delle piccole sponsorizzazioni, tant'è vero che l'articolo 7 riprende la possibilità di migliorare le agevolazioni fiscali previste dalla finanziaria del che erano state approvate anch'esse all'unanimità su proposta dell'allora sottosegretario Pescante, in connessione ad un emendamento presentato dal sottoscritto e dall'attuale onorevole Giovanni Lolli. Il sottosegretario Crimi si è già espresso favorevolmente in Commissione, sottolineando tra l'altro, come dice l'indagine del CONI, come oggi vi sia la preoccupazione di un grande abbandono da parte dello sport della fascia dai 15 ai 17 anni. che vi sia, all'indomani di un grande successo per lo sport italiano come il trionfo dell'Inter nella Champions League, la volontà di valorizzare il volontariato nello sport di base, anche perché questo provvedimento

Signora Presidente, io non troverei un'espressione, un concetto più adatti per motivare la richiesta di modifica dell'ordine dei lavori della settimana prossima,

il Governo deve fare i conti con un quadro economico e finanziario assolutamente preoccupanti. Per questa ragione, credo sia questo il momento degli interventi di riforma veri, di carattere strutturale, continuativo, e non di interventi più o meno palliativi che oggi servono semplicemente per mettere la polvere sotto il tappeto. Per questa ragione chiedo che la prossima settimana si possa discutere qui in Aula del tema relativo all'amministrazione straordinaria per le imprese in crisi, crisi, vale a dire uno strumento o un istituto che serve al buon funzionamento dei mercati, in modo particolare del mercato interno. Prima di soffermarmi un attimo sul tema dell'amministrazione straordinaria, vorrei insistere sulla necessità di provvedimenti di carattere continuativo e porto un esempio, tenuto anche conto di quanto esce riferimento alla manovra che verrà presentata tra pochi giorni all'attenzione della nostra Aula. Faccio riferimento ad alcuni provvedimenti un po' farraginosi

Sarebbe invece importante che a questo istituto venisse restituita la sua funzione di gestione della crisi di impresa (non necessariamente della liquidazione), per le imprese che hanno una soglia superiore ai 200 o ai 500...

che la prossima settimana si finisca in una discussione che non può far altro che acutizzare la crisi nel rapporto fra la politica e il Paese, tra noi e i

si conviene sul fatto che questo Paese, e quindi questa Camera, abbia ben altre priorità da affrontare. Si conviene anche sul fatto che questa

a soluzioni più mature, in grado di garantire l'azione a tutela della legalità e di contrasto alla criminalità, salvaguardando al tempo stesso i diritti fondamentali dei cittadini.

dal non utilizzo delle migliori tecnologie, dalla mancata adozione di strumenti in grado di prevenire situazioni di disastro. Per questo motivo chiediamo che venga discusso il disegno di legge n. 1920, che propone modifiche al decreto legislativo n. 625 del 1996, non solo determinando una diversa modalità di definizione dei canoni per la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ma anche mettendo in campo azioni a tutela dell'ambiente, attraverso l'uso delle migliori tecnologie disponibili, e inducendo in questo modo gli operatori di idrocarburi a rispettare modalità che consentano di salvaguardare l'ambiente e di preservare la salute dei cittadini. Il territorio nazionale presenta livelli di fragilità

per una ragione molto semplice: il disegno di legge sulle intercettazioni, oltre a creare un *vulnus* per la nostra democrazia, oltre a mettere in difficoltà i magistrati nell'opera di perseguimento di reati importanti, toglie spazio ai provvedimenti che sono urgenti per davvero, che sono quelli indicati

della banda larga e alla diffusione del *software* libero. Il motivo è molto semplice: la crisi economica che in questi due anni ha devastato l'Europa e il mondo intero è stata affrontata nei grandi Paesi industriali prevedendo grandi investimenti sulle nuove tecnologie della comunicazione. In tutti i Paesi, con una sola poco lodevole eccezione: l'Italia. L'Italia è rimasta al palo e lo è rimasta con il piano del vice ministro Romani che ha promesso, più di un anno fa, un programma di 800 milioni di euro per la banda larga. Finora non è stato speso praticamente nulla e quel piano è ormai nei cassetti, è lettera è lettera morta, un piano che, a detta dello stesso Governo, avrebbe generato almeno 50.000 posti di lavoro nel nostro Paese, con benefici enormi per la competitività del nostro sistema produttivo, con la possibilità davvero di far decollare una pubblica amministrazione di qualità, capace di rispondere con la digitalizzazione al nuovo dialogo tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Di più. In questi giorni il professor Mario Monti nella relazione per il presidente Barroso ha individuato nel mercato unico digitale uno degli obiettivi strategici di fondo per il rilancio economico dell'Europa, per il rilancio delle stesse istituzioni europee, perché in quel mercato unico digitale ci sta gran parte dei nuovi motori per lo sviluppo del nostro continente.

Mi permetto però di aggiungere una considerazione più specifica riguardo una mia spiccata sensibilità verso una vicenda che proprio questo calendario parlamentare consente di riproporre all'attenzione del Paese.

che le ragioni di custodia cautelare fossero determinate dal fatto che nel corso degli interrogatori non emergesse alcun elemento per interrompere tale custodia cautelare. Questa concezione dell'istituto dell'interrogatorio è cinica, odiosa e antitetica al dettato della nostra Costituzione. A questo si aggiunge che proprio in connessione con questa discussione del Senato, non più tardi di qualche sera fa è comparso televisivamente uno dei magistrati procedenti. Non ne faccio il nome perché non è mio costume, neanche negli atti di sindacato ispettivo. Si trattava di un magistrato della procura della Direzione distrettuale antimafia, il quale ha detto che questa concezione della custodia cautelare era corroborata dal decisivo apporto

possa trarre da questo calendario parlamentare una ragione per rispolverare dalle sovrintendenze archeologiche l'istituto dell'esercizio della responsabilità disciplinare. *(Commenti del senatore

ma se permette, come senatore della maggioranza, la ringrazio anche di avere altrettanto efficacemente garantito la libertà di interruzione su volgarità che non recepisco. LUSI *(PD)*. Le volgarità sono

Maritati, quando si dà la parola è buona prassi, quando possibile, alternare interventi dei due schieramenti, come lei

ciascuno di noi ne ha avuti tre a disposizione, fondamentalmente per dimostrare due cose, che mi permetto di sintetizzare. La prima è questo Senato non sta svolgendo la propria funzione. Sostanzialmente, questo ramo del Parlamento si trova in una condizione di commissariamento. del Parlamento è commissariato dal Governo, il quale, di intesa con le rispettive Presidenze - e allargo il discorso anche alla Camera dei deputati permette il transito esclusivo di provvedimenti di origine governativa ed il regolare blocco di di tutti i provvedimenti di iniziativa parlamentare. Dunque diciamo a voce alta, per chi ha la voce più alta della mia, che ci troviamo in una condizione di sospensione di un esercizio democratico.

la nostra completa, ancorché inquieta, conoscenza della realtà: il cosiddetto provvedimento sulle intercettazioni è finalizzato, a nostro giudizio, a domare definitivamente ciò che è rimasto della stampa libera e a sfinire una volta per tutte l'ordinamento giudiziario, in modo tale che sotto lo stivale del potere governativo quest'ultimo possa soccombere. Così facendo, signora Presidente, il Governo e la maggioranza stanno assecondando le aspettative di quella parte del loro blocco sociale di riferimento che ora sarà costituita, oltre che da evasori e da condonati, anche da impuniti.

La percezione di questa lontananza continua ad essere suffragata dai comportamenti posti in essere all'interno di quest'Aula.

seguente tema: in genere il costo deve essere commisurato ad un valore e il valore che noi esprimiamo nei confronti del Paese sul lavoro che compiamo non corrisponde al costo stesso. Non corrisponde al costo perché

siamo lenti nel dare le risposte correlate ai compiti che ci sono assegnati rispetto alla velocità con la quale si muove la vita reale.

reale, ci dobbiamo preparare a comunicare al Paese una manovra che determinerà sicuramente una accentuazione dell'immobilismo dell'Italia. Credo che la modifica del calendario ci consenta di dimostrare due fatti. In primo luogo, esiste un valore nel lavoro dei parlamentari l'elenco delle proposte che sono state richiamate e che devono essere discusse in questa Aula dimostrano che il lavoro dei parlamentari esiste e che con esso potremo riuscire anche a

La seconda dimostrazione è quella del valore

molto apprezzabili. Mostra che i senatori hanno lavorato in questo periodo, e che quelli dell'opposizione hanno nel cassetto - purtroppo nel cassetto - proposte significative nei

provvedimenti, ce ne sono alcuni che riguardano proprio l'aspetto della rassicurazione. In un momento di crisi, la paura, l'inquietudine, l'incertezza aumenta; noi abbiamo presentato diversi provvedimenti, in particolare uno che riguarda i cosiddetti ammortizzatori sociali, che da tanto tempo sollecitiamo. È molto maturo, ma non è arrivato in Aula e vi dovrebbe giungere, perché questo darebbe sicurezza

cominciato a discutere, ma che dovrebbe essere prioritario in questo momento, riguarda il sostegno dell'occupazione (in realtà si tratta di più di un provvedimento), perché dobbiamo pensare a come riprenderci da questa crisi e solo sostenendo il lavoro, che invece è depresso e ridotto, possiamo avere una ripresa che non sia priva di lavoro. Al riguardo abbiamo fatto proposte; qualcuno ha già parlato delle proposte per il lavoro femminile, ma in realtà pensiamo che la politica del lavoro debba occuparsi...

Signora Presidente, anch'io farò una proposta di modifica del calendario. Voglio in premessa richiamare un auspicio, auspicio, ossia che domani si possa raccontare del lavoro di questa mattina dell'opposizione, del Partito Democratico in particolare, nell'Aula del Senato non come di una ennesima occasione di allungamento dei tempi, una forma di ostruzionismo (come si può dire banalmente), quanto del tentativo di dimostrare al Paese che c'è una parte del Parlamento che vuole occuparsi dei problemi veri degli italiani, dei cittadini, delle imprese, dei territori. L'elenco, lungo, che abbiamo fatto qui, a cui io unirò un ennesimo capitolo, dimostra come il Paese sia impegnato in queste settimane e in questi giorni a pensare ad altro che non al tema che invece la protervia di una maggioranza e del Governo vorrebbe imporre con un ordine del giorno mutato in corso dei lavori. Sono qui a proporre che le prossime sedute dell'Aula del Senato vengano impiegate in una informativa urgente dell'attuale titolare del Ministero dello sviluppo economico, che - come sappiamo - è gestito *ad interim* dal presidente Berlusconi (un *interim* che doveva durare pochi giorni, ma che ormai va verso il mese), su una vicenda che interessa tanto gli italiani, ossia il ritorno all'energia nucleare nel nostro Paese. Vi è nel Paese una grande confusione; sono molti i territori in allarme rispetto alle ipotesi che girano, non accreditate, sull'individuazione dei siti. Vi è un grande contrasto istituzionale tra gran parte delle Regioni italiane e lo stesso Governo, giunto finanche alla Corte costituzionale. Non è nostra intenzione riaprire qui la discussione di merito, né tornare ad uno scontro quasi ideologico sul merito delle questioni. Vorremmo però assieme al Paese reclamare in quest'Aula, alla presenza del Ministro dello sviluppo economico e del Presidente del Consiglio, certezze per il Paese, certezze sulle norme, sulle procedure, sugli strumenti di garanzia. Sono passati dieci mesi dall'approvazione della legge delega, due mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo sui criteri per i siti; entro febbraio il CIPE avrebbe dovuto deliberare - e non l'ha fatto - criteri per la costituzione dei consorzi di imprese; entro il 23 maggio - e non c'è ancora - avrebbe dovuto essere emanato un decreto ministeriale sulla certificazione dei siti. Siamo nella più grande confusione. L'Agenzia per la sicurezza nucleare è in alto mare, non c'è ancora lo statuto, non ci sono i regolamenti attuativi, non ci sono le norme. Appena qualche settimana fa l'allora ministro Scajola parlava del 2013 per il primo cantiere aperto; qualche settimana fa il sottosegretario Saglia, più realisticamente, ha parlato del 2013 come data per la localizzazione dei siti. Ce n'è abbastanza perché il Senato torni ad occuparsene e faccia uscire...

di modificare il calendario e di tornare ad occuparci dei problemi reali del Paese e delle nostre comunità. Ce n'è una in particolare, che non è una piccola comunità, ma è la città di Roma, di Roma, la cui amministrazione ancora a fine maggio non ha approvato il bilancio, né ha presentato una bozza di bilancio.

(le cui dimensioni cambiano a seconda delle dichiarazioni e dei manifesti che appaiono in città), venga urgentemente a riferire in Aula su cosa sta succedendo. Sui giornali di oggi, a differenza di quanto diceva il *premier* e qualcuna delle persone che in genere riferiscono il suo parere, per i cittadini di Roma è previsto un consistente prelievo fiscale, con l'aumento delle aliquote IRPEF, con una serie di balzelli e di pedaggi e con una misura che va a pesare fortemente sull'economia della città di Roma, che per il 12 per cento è legata alle presenze turistiche, relativa ad una tassa di soggiorno di proporzioni anche piuttosto consistenti. Tutte cose, tra l'altro, che smentiscono quello che si era detto durante la recente campagna elettorale, come se le cose che si dicono non abbiano senso. Ripeto: la città non ha il bilancio e credo che chi ha fatto l'amministratore sappia cosa vuol dire questo in termini di programmazione, investimenti e lavoro. Viene annunciata un'ipotesi per fine luglio, quindi sostanzialmente tutto il 2010 rischia di passare, in un Comune così importante, senza lo strumento principale della politica amministrativa di una città o di un Comune, che è appunto il bilancio. Ecco perché chiediamo che si venga qui a prendere atto della vicenda e a raccontare ai cittadini di Roma e agli italiani, che devono in qualche modo essere partecipi di tale situazione, della quale quale il Parlamento e il Governo in carica si sono occupati una decina di volte, qual è la verità e qual è la presa di coscienza anche in questo caso. Assistiamo costantemente a dichiarazioni, smentite poi dalla faccia del sindaco, che esce piuttosto scuro dai colloqui a Palazzo Chigi. Chiediamo che vi sia una discussione su questo e che non si cerchi ogni volta di accantonare i problemi reali del Paese, prendendo a pretesto i problemi di qualche singolo che ha necessità di coprire intercettazioni imbarazzanti. Presidente, onorevoli colleghi, come evitare, quando torniamo a casa alla fine di questa settimana di lavori parlamentari, il sentimento di vergogna che provoca il riferire ai propri cittadini che non ci si è occupati di nulla, purtroppo, di quello che morde la carne delle situazioni di maggiore difficoltà del nostro Paese? È questa la ragione per la quale vi chiedo di votare, nel sovvertire il calendario approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, per discutere immediatamente di un caso che rischia di essere dimenticato tra le tante crisi italiane, quello racchiuso in una mozione di cui sono primo firmatario. Si tratta del caso della Eurallumina Srl, una società di proprietà di una grande multinazionale russa, l'unica produttrice della materia da cui si fa l'alluminio, una materia strategica, importante nel Paese e in Europa, il cui unico luogo di produzione del Mediterraneo, in Sardegna, a Portovesme, da oltre un anno è chiuso. È chiuso per una crisi di mercato, ma anche per una strategia di delocalizzazione da parte delle grandi società che producono nel mondo in questo settore. C'è qualcosa che non torna nella gestione della crisi di Eurallumina Srl da parte del Governo. Vedete, colleghi, noi con la Russia trattiamo grandi investimenti, interventi strategici, alleanze militari; trattiamo anche la cessione del pacchetto di maggioranza di proprietà del Milan nelle residenze private del *Premier* e nei dintorni, non trattiamo - ci sembra di capire - il tema, che è di politica economica ma anche di geopolitica, di come persuadere uno dei più grandi gruppi russi a tornare ad aprire l'unico impianto mediterraneo che avrebbe già oggi la convenienza a riaprire. C'è qualcosa che non va. C'è una crisi di cui si deve occupare il Parlamento e non lo fa perché è impegnato a discutere di intercettazioni. Ma vi è una crisi del sistema produttivo di cui deve occuparsi quotidianamente il Governo. Da 20 giorni - è stato già ricordato - il Ministero dello sviluppo economico è affidato all'*interim* del Presidente del Consiglio. Ci sono centinaia di tavoli di crisi aziendale gestiti nel Ministero dello sviluppo economico affidati a pur volenterosi funzionari, ma senza la guida politica di un Ministro in carica. Il Paese, il nostro sistema produttivo, la crisi economica di questo Paese non sono in mani salde, colleghi senatori, ed il momento non lo consente. Torniamo ad occuparci delle cose vere...

sulle intercettazioni non sia posto all'esame dell'Aula il prossimo 31 maggio e che venga invece posto all'attenzione della competente Commissione giustizia, propongo all'attenzione della Presidenza e dei colleghi tutti una proposta di modifica al calendario. venga inserito nel calendario dei lavori dell'Aula, a partire dalla prima seduta della prossima settimana, l'esame della mozione n. 181 concernente la predisposizione di un Piano per l'area industriale della difesa, Un piano tanto più necessario in questa straordinaria situazione di difficoltà del nostro sistema-Paese, un piano a difesa dell'occupazione nel settore in grado di rilanciare un comparto essenziale per il nostro sistema militare in termini di efficienza e qualità dei mezzi impiegati. Infatti, un pieno rilancio dell'area industriale della difesa è una delle chiavi per una razionalizzazione dello stesso modello di difesa, che non può avvenire, come fatto fino ad oggi, unicamente con i tagli lineari alla spesa di funzionamento e di esercizio. D'altra parte, signora Presidente, la crisi e le difficoltà della nostra economia richiamano l'esigenza di interventi strutturali ed anche questo settore può essere il luogo per realizzare azioni efficaci in tal senso. Un contributo anche dall'area industriale della difesa, quindi, è possibile per rilanciare la crescita e per migliorare la qualità della nostra spesa pubblica. È nota la necessità, spesso da noi segnalata, di una radicale revisione dell'insieme di capitoli e programmi concernenti la spesa per la difesa in un quadro di reale e concreto taglio degli sprechi e di una migliore utilizzazione delle risorse a disposizione e da impiegare. Anche per queste ragioni sottolineo l'importanza dell'argomento proposto che, seppur parziale rispetto al complesso della manovra economica e finanziaria che attende il nostro esame, risulta in ogni caso utile al complesso dei necessari interventi da effettuare per contribuire al superamento della crisi e per migliorare la nostra finanza pubblica. *(Applausi *(PD)*. C'è una necessità di intervenire sul tema delle intercettazioni? Credo di sì. C'è questa esigenza, ma non riteniamo che questa possa essere elevata al rango di priorità. Una legge che, se attuata, se varata così come uscita dalla Commissione giustizia, avrebbe soltanto come risultato di censurare - sì, dico censurare - per un periodo di anni la stampa italiana e limiterebbe gravemente la capacità di risposta repressiva giudiziaria dello Stato contro la criminalità di ogni tipo. Tutta la fretta che sta caratterizzando il comportamento della maggioranza e del Governo non è quindi espressione di una sensibilità democratica, che è cosa diversa peraltro - del tutto diversa - dall'idea espressa sorprendentemente dal senatore Quagliariello questa mattina, al quale risponderò a tempo debito cercando veramente, con tutte le mie capacità, di spiegargli qual è la differenza tra il sistema dittatoriale e una invasività di un organo di spionaggio interno, da un lato, e le disposizioni legittimamente impartite da un organo giudiziario in un sistema democratico. Dicevo: no. La fretta di La fretta di discutere il disegno di legge sulle intercettazioni non è espressione di una sensibilità democratica. È piuttosto l'espressione di un inconfessabile quanto evidente interesse di persone o gruppi che hanno una gran paura di essere smascherati nelle nefandezze che vanno sistematicamente consumando ai danni della società onesta che il Parlamento dovrebbe sapere ben tutelare.

Perché non si dà a questo disegno di legge priorità rispetto a quello sulle intercettazioni? È su queste scelte, senatore Quagliariello, che si può offrire la prova del proprio DNA, democratico o meno. È per questo che chiedo che il Senato nelle prossime giornate di lunedì e martedì discuta e vari questo disegno di legge. Che vergogna! Che danno per l'Italia per questi ritardi!

solo apparentemente limitato - di opacità, di difetto di trasparenza di comportamenti pubblici (in questo caso quelli del Governo greco nei mesi passati), a noi sembra che sia totalmente fuori luogo la priorità assoluta con cui il Governo italiano vuole imporre al Senato l'esame di un disegno di legge che sostanzialmente muove in direzione di una minore trasparenza complessiva delle nostre istituzioni e della nostra società civile. Noi siamo dell'opinione opposta, ci sembra cioè che in questo momento si debbano mettere prioritariamente all'ordine del giorno misure di trasparenza totale.

a firma mia, della presidente Finocchiaro e di numerosi altri senatori del Partito Democratico e radicali, mirato all'istituzione di una anagrafe degli eletti direttamente accessibile *on line,* per la visibilità dei redditi e dei patrimoni

presidente Finocchiaro e dei senatori Zanda, Morando, Nerozzi, Treu e Vimercati, in materia di trasparenza e possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza.

Signor Presidente, anch'io voglio chiedere la modifica del calendario d'Aula perché vorrei

È un problema sociale e pertanto devono essere coinvolti enti ed istituzioni operanti nell'ambito sociosanitario. L'informazione e la prevenzione in questo caso sono importanti, ma anche la cura e la riabilitazione. Le cronache sovente ci riportano aspetti drammatici di cui sono protagonisti i grandi obesi, ad esempio la difficoltà di eseguire una problemi di mobilità e di attrezzatura, nei luoghi pubblici ma, soprattutto, nei luoghi di ricovero, cioè negli ospedali. Va quindi da sé la richiesta dell'abbattimento delle barriere architettoniche per consentire un'adeguata vita sociale

però voglio far notare che questo è stato esteso anche alle categorie protette, perciò anche ai disabili; si potevano usare le graduatorie esistenti, sarebbe stato un bel segno di attenzione per i più deboli. Noi del Partito Democaticio questo non lo avremmo mai fatto.

che prima di discutere il disegno di legge sulle intercettazioni si programmi nei nostri lavori la discussione di un altro disegno di legge, che è essenziale, anche ai fini di intervenire, se mai si vorrà farlo, sulla questione delle intercettazioni. Infatti, sin da quando è iniziato il dibattito (ormai più di un anno fa, anzi, forse sin dall'inizio della legislatura) da più parti si è sottolineato che un intervento sulle intercettazioni, così come vorrebbe fare il Governo nelle varie formulazioni che si sono susseguite in questi mesi, colpirebbe, tra l'altro, una fattispecie di reati

che possono ottenere dal traffico della droga. Se noi non interveniamo sul disegno di legge che prevede

nel definire come comportamenti criminosi i reati ambientali da inserire nel codice penale, avremo il paradosso che poi, intervenendo soltanto sul fronte intercettazioni, impediremo alla magistratura di perseguire quella tipologia di reati lasciando in libertà mafiosi, criminali e camorristi che sul

Signor Presidente, sono a chiederle anch'io di modificare il calendario dei lavori dell'Aula. Presidente, noi siamo reduci da una settimana in cui sul fronte della televisione pubblica è successo di tutto: conduttori che litigano usando le proprie trasmissioni per discutere dei loro contratti milionari, rimproverandosi l'un l'altro di guadagnare troppo. Abbiamo all'attenzione dell'8a Commissione del Senato - è questo il cuore del mio ragionamento - una proposta di cui è prima firmataria la presidente Finocchiaro, ma sullo stesso argomento insistono progetti di legge anche di colleghi del centrodestra, tesi a riformare la *governance* (una brutta parola inglese) della RAI, cioè a riformare criteri e natura del consiglio di amministrazione di tale ente. Lo sanno i colleghi che mentre dilaga, a volte giustamente - qualche volta ingiustamente - una forte campagna contro quello che guadagnano i parlamentari, il loro ruolo e la casta (sono anni che va avanti, complici spesso anche la televisione e certi conduttori), noi, in virtù della legge Gasparri, abbiamo un consiglio di amministrazione della RAI i cui nove componenti percepiscono compensi non a gettone, come avviene per i consigli di amministrazione di tutte le aziende del mondo, pubbliche o private che siano, e che sono superiori a quello dei parlamentari in carica? Lo sapete che il direttore generale della RAI guadagna cinque-sei volte più di un parlamentare? Lo sanno i colleghi che anche il presidente della RAI, figura di garanzia e con scarsi poteri di direzione manageriale, manageriale, guadagna cinque-sei volte più di un parlamentare? Allora, mentre questo Governo, Presidente - e mi avvio alla conclusione - sottopone al Paese una manovra lacrime e sangue, forse sarebbe ora che il Parlamento desse un segnale. Bastano due giorni di lavoro in Commissione per trovare un accordo e riformare i criteri e la natura del consiglio d'amministrazione. Oltre a fare una cosa giusta in sé e a consentire alla RAI di essere un'azienda normale e non un bottino di guerra di maggioranze che si alternano, forse produrremmo anche dei risparmi più significativi delle tante chiacchiere sui parlamentari. *(Applausi Signor Presidente, sono intervenuti molti colleghi del Partito Democratico, alcuni ponendo anche questioni connesse al tema principale che oggi preoccupa gli italiani, che è il tema della manovra economica, il tema dei sacrifici che devono essere fatti, il tema di come affrontare questo momento difficile pensando di incidere su chi ha effettivamente i privilegi e di non rendere la vita impossibile a chi ha difficoltà, molti altri molti altri portando ulteriori argomenti interessanti, ricordando comunque che questo provvedimento sulle intercettazioni non è così urgente. È abbastanza grave che in questo Senato e, complessivamente, in questo Parlamento, molte delle ore del nostro lavoro siano state spese su provvedimenti legati alla questione giudiziaria, ma non per il miglioramento del sistema giustizia, di cui ci sarebbe bisogno, bensì per questioni specifiche che riguardavano i processi

il lavoro di quest'Aula. Ultimamente siamo stati presi di mira sui giornali per la mancanza di lavoro in Senato, anche con statistiche che poi non corrispondono al vero, perché non viene valutato il lavoro delle Commissioni; ma,

È una piccola questione, che però se tocca a qualcuno in particolare diventa grande e pesante. Cito questo caso, perché sul provvedimento il ministro della difesa La Russa in due interviste sui giornali e in numerose dichiarazioni in televisione ha già detto che è d'accordo sul fatto che non vi siano limitazioni. Quindi, basterebbero pochi minuti di lavoro per eliminare quel che può essere un possibile fattore di ingiustizia. Anche questo non viene fatto perché dobbiamo occuparci di altro. Ho voluto cominciare dalla questione economica perché ritengo che sia davvero centrale ma passo anche per questioni che possono sembrare minimali, ma che potrebbero mettere a posto alcune storture esistenti, per dire che

Signor Presidente, vorrei chiedere, a modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea proposto dal presidente Schifani e dalla Conferenza dei Capigruppo a maggioranza, che la prossima settimana quest'Aula possa ascoltare una relazione del Governo sulla situazione delle Regioni nelle quali il piano di rientro della spesa sanitaria appare inadeguato e insufficiente, tanto è vero che la scorsa settimana il Consiglio dei ministri ha deciso di sospendere l'erogazione dei contributi nazionali prelevati dai fondi FAS a quelle Regioni che non hanno adempiuto agli impegni sottoscritti nella stipula dei piani di rientro. Si parla del Lazio, della Campania, della Calabria e di altre Regioni ancora. Forse quest'Aula avrebbe diritto a sapere cosa sta succedendo, e immagino la faccia sorpresa della giovane e simpatica presidente della Regione Lazio Polverini, quando ha scoperto che il Consiglio dei ministri ha deciso che quella ristrutturazione della rete ospedaliera per oltre 3.000 posti letto è uno degli impegni che devono essere rispettati imponendole, con il taglio dei finanziamenti, di presentare entro la fine

fatto che il Popolo della Libertà non avrebbe consentito il taglio di nessun posto letto nella Regione Lazio. Cosa è cambiato? Davvero, colleghi, cosa sta cambiando? Forse è bene che il Governo ce lo spieghi. Il commissario del Governo, che non era peraltro neanche presidente della Regione Lazio, lo stimatissimo professor Elio Guzzanti, dopo essere stato presidente per cinque mesi, non ha presentato il piano di riconversione della rete ospedaliera. Anche per questa ragione, la Regione Lazio adesso è costretta ad aumentare le tasse ai propri cittadini - l'IRAP e l'IRPEF - e quelli che vivono nel Comune di Roma hanno la fortuna, come ricordava il collega Milano, di non avere neanche il bilancio comunale e di avere una manovra, approvata ieri, nella quale si dice che bisogna aumentare anche la sovrattassa IRPEF comunale. Cosa sta accadendo? Io penso che sarebbe utile, colleghi, se il Governo, se il cattivo ministro Tremonti venisse a spiegare cosa sta succedendo nel rapporto con le Regioni ed in particolare con la Regione Lazio e il Comune di Roma.

È questa forse la dimostrazione più lampante delle potenzialità inespresse nelle Aule parlamentari: un Parlamento che mai come in questa legislatura è mortificato e dileggiato, è stato ricordato anche dagli interventi prima del mio, a partire proprio dalla calendarizzazione dei provvedimenti all'esame dell'Aula, frutto, come in questo caso, del provvedimento sulle intercettazioni da noi avversato perché rispondente a logiche estranee alle necessità reali del Paese e rispondenti agli interessi dei soliti noti. Così facendo, viene mortificata la dignità residua delle massime istituzioni del Paese, in un gioco ormai allo sfascio, incurante per di più della grave situazione che il Paese sta attraversando.

da me presentata insieme ad altri 35 colleghi il 23 aprile 2009 ma ancora di particolare e stringente attualità, riguardante il comparto del trasporto aereo. Profonde e significative novità sono infatti intervenute nel settore a partire dal 13 gennaio 2009, data in cui è avvenuto il passaggio di consegna ufficiale della compagnia di bandiera, da parte del commissario liquidatore di Alitalia S.p.A., alla compagnia aerea italiana, la cosiddetta CAI. Tutti noi viaggiamo sovente in aereo e vediamo materialmente come il passaggio dell'ex compagnia di bandiera alla CAI è stato finora contrassegnato da pesanti perdite economico-finanziarie non solo per il bilancio dello Stato, ma anche per migliaia di cittadini che avevano investito i propri risparmi in Alitalia, la cui quantificazione è ancora incerta. Ma particolarmente oneroso è stato il costo sociale dell'operazione sul versante occupazionale. La CAI, infatti, deciso di assumere la somma dell'operativo Alitalia-Air One ridotto del 30 per cento. Il totale del personale dell'ex Alitalia messo in cassa integrazione, tra piloti, assistenti di volo e personale di terra, è pari a 7.000 dipendenti. La CAI nel suo piano industriale ha previsto il raggiungimento del *break-even* entro il 2010, fissando al 65 per cento il livello medio del coefficiente di occupazione degli aerei. Sappiamo che quegli obiettivi, al di là dei toni trionfalistici usati...

C'è una manovra di cui non si sa niente e ciò che sappiamo non ci piace, c'è una manovra che peserà pesantemente sulle persone più deboli di questo Paese e soprattutto sul lavoro dipendente. Proprio in una fase di questo genere, la coesione sociale è importante, decisiva. Noi abbiamo superato le crisi di questo Paese, penso al 1993 e anche a situazioni precedenti, solo lavorando sulla coesione sociale, lavorando sull'unità di tutte le forze sociali.

e la rappresentanza sindacale - provare ad unire ciò che voi volete dividere, è necessario dare la possibilità alle lavoratrici e ai lavoratori di poter conoscere e decidere ciò che avverrà, poter in qualche modo almeno dire il proprio parere; è necessario, raccogliendo l'accordo unitario CGIL-CISL-UIL dare un quadro che possa permettere di avere

i più deboli, inventando sindacati di comodo, di condominio o di piccolo territorio come avete fatto nell'ultima legge. Non si supera in questo modo, ma coinvolgendo l'insieme delle forze sociali, da quelle più rappresentative, da quelle che hanno la fiducia, il peso, gli iscritti e i voti dei lavoratori e aiutando queste forze sociali ad unirsi e non a dividere come fate quotidianamente con incontri di notte nei sottoscala e nelle cantine.

la priorità assoluta dovrebbe averla la presenza del ministro Tremonti in quest'Aula lunedì prossimo per una discussione di inquadramento delle tematiche generali di carattere economico-finanziario su cui contestualizzare e poter meglio valutare le misure definite con la manovra sui conti pubblici di cui si è deciso in questi giorni. Con l'occasione, il ministro Tremonti potrebbe dare conto al Parlamento degli esiti che ha dato complessivamente, con tutti i dettagli utili ad esprimere analisi e giudizi, il discusso provvedimento sullo scudo fiscale, come peraltro lo impegna a fare una norma approvata con il decreto Ma ci sono anche provvedimenti di portata meno generale che hanno sicuramente più urgenza e necessità di venire alla discussione in quest'Aula rispetto al controverso disegno di legge sulle intercettazioni. Ad esempio, l'annosa questione dei crediti vantati da imprese italiane nei confronti della Jamahiriya libica. Si tratta di una questione aperta ormai da almeno tre legislature. Ma ora il relatore, senatore Mura, dopo aver fatto un'importante lavoro di sintesi dei vari disegni di legge proposti (tra cui uno anche a mia firma), ha proposto un testo unificato che ha ottenuto l'adesione di tutti in Commissione finanze. Il provvedimento non presenta neppure problemi sotto il profilo della copertura finanziaria, perché è ampiamente garantito dal complesso dei trasferimenti previsti nell'ambito del Trattato di amicizia tra l'Italia e la Libia, e fissa l'importo delle somme da rimborsare, con un'ulteriore penalizzazione per le imprese italiane, a 450 milioni di euro, cioè l'importo che anche la parte libica, come ci disse il ministro Frattini in quest'Aula nel settembre del 2008 e poi successivamente in Commissione, riconosce essere richiesta legittima da parte delle imprese interessate. Dunque, si può fare. E l'urgenza è dettata dal lungo tempo ormai trascorso, dai già enormi danni economici subiti dalle imprese, dalle ulteriori difficoltà generate dalla crisi economica e dalle strette creditizie. Se noi lo approvassimo lunedì o martedì - e sarebbe possibile - la Camera dei deputati potrebbe assumere l'atto prima dell'estate. Sarebbe un modo minimo di testimoniare e di esprimere giustizia riparatrice verso le tante imprese interessate e, soprattutto, la dimostrazione

mesi abbiamo imparato ad apprezzare il lavoro di alcuni che non la pensano come noi, ma che lavorano alacremente. Però voi obbedite ad una richiesta ideologica: vi si chiede di stare in Aula, di tenere il posto, di votare anche provvedimenti su cui non siete d'accordo. La disciplina di Gruppo è importante certe volte, ma per quanto tempo potete reprimere la possibilità di diventare finalmente una destra europea e normale: una destra europea e normale che possa vincere in questo Paese non solo con il populismo e che non sia schiava di un padrone solo? Questa nostra riflessione, quindi, non è inutile. Serve per dialogare con voi perché sappiamo che sentite che questo provvedimento è sbagliato sbagliato e che, soprattutto, mette in difficoltà voi perché dimostra che non siete in grado di modificare un lavoro che avete fatto strutturalmente. In ultimo,

come è finita la vicenda del nostro impegno per l'Abruzzo. Anch'io, signor Presidente, credo che il disegno di legge sulle intercettazioni rivesta un'urgenza molto inferiore rispetto ad altri provvedimenti. Chiedo, quindi, che il calendario dei lavori sia modificato per attribuire priorità ad un atto che il Parlamento dovrebbe esaminare in tempi brevi perché attiene alla salvaguardia dei diritti umani, impegno sempre esaltato dal nostro Paese. Mi riferisco alla ratifica di un trattato internazionale che quelle finalità umanitarie persegue proprio nelle circostanze in cui esse sono maggiormente in pericolo, cioè nei conflitti armati. Il 28 maggio 2008, all'inizio della legislatura, il Senato impegnava il Governo con un ordine del giorno a sostenere il Trattato per la messa al bando delle *cluster bomb* (le bombe a grappolo); un trattato concepito, elaborato e promosso per salvaguardare l'incolumità di coloro che sono le vittime più frequenti di quegli ordigni, ossia la popolazione e in particolare i bambini. Ebbene, dopo due anni - oggi siamo al 26 maggio - il Parlamento italiano non ha ancora ratificato quel Trattato, e ciò in presenza di scadenze ormai vicinissime, quale la sua entrata in vigore, prevista per il 1° agosto del corrente anno, anno, e soprattutto nonostante il fatto che l'impiego di quegli ordigni tuttora colpisca degli innocenti. Credo quindi che il Parlamento non possa dilazionare ulteriormente la sua decisione al riguardo, e soprattutto che l'Italia non possa risultare ancora assente tra le Nazioni che già hanno compiuto questo passo determinante. Chiedo pertanto che alla ratifica di quel Trattato venga data nei nostri lavori la massima priorità. *(Applausi dal Signor Presidente, colleghi, sarebbero diverse le questioni da mettere all'ordine del giorno, alcune delle quali da tempo rinviate. Mi si potrà dire - per esempio - che la ratifica della Convenzione europea per gli animali da affezione potrà essere prestissimo calendarizzata, ma questo succede da lungo tempo e ancora non è avvenuto, a differenza della Camera che già a novembre ha ratificato questo atto. Non credo si tratti solamente di un disguido o di una serie di coincidenze. Ho l'impressione che ci sia la volontà di non arrivare in fondo ad una pratica importante che vede l'Italia diventare finalmente maggiorenne e quindi assumersi responsabilità su questioni molto importanti.

Allora, chiediamo che sul tema del randagismo, su un tema come questo che deve essere controllato, su una nuova forma di legislazione importante che riguardi gli animali da affezione, ci sia maggiore attenzione. Anche quando riusciamo ad ottenere proposte di leggi *bipartisan*, anche quando abbiamo mozioni *bipartisan*, poi però non si va avanti. La settimana scorsa ho assistito ad una conferenza stampa della sottosegretaria Martini proprio sulla tutela degli animali da affezione e sul randagismo: un bellissimo video e una bellissima Sottosegretaria, ma non vi è stato alcun momento di confronto su temi che noi siamo in grado di affrontare e che vogliamo discutere insieme. Reputo assolutamente importante che su tali questioni si presti una maggiore attenzione, anche perché, quando si parla di crisi e di povertà, si deve sapere - credo che qui si sappia - che molto spesso alcuni animali da affezione sono l'unica ed ultima compagnia di tante solitudini. Questa, quindi, è una questione che ci appartiene in modo importante. Un animale da compagnia vive in una famiglia su quattro. Parlare di vivisezione e di leggi che riguardano la medicina veterinaria convenzionata vuol dire rispondere ad esigenze del Paese, alle famiglie del Paese, alle povertà dei nostri anziani e anziane. Signor Presidente, le chiedo una modifica del calendario presentato dal Presidente Schifani ed approvato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo. In particolare, le chiedo di espungere il disegno di legge sulle intercettazioni calendarizzato per lunedì prossimo ed inserire al posto di questo argomento la mozione n. 185, di cui sono primo firmataria, che riguarda il tema della scuola. È stato più volte rilevato da vari colleghi del Gruppo come le priorità per il nostro intervento e per le nostre votazioni attengono ai temi di rilevanza economica, sociale, culturale del Paese. Io credo che nel nostro Paese si stia verificando una vera e propria emergenza educativa. Accanto alla grande emergenza di carattere occupazionale ed economico vedo una profonda difficoltà di tutte le strutture educative. E questo è fortemente condizionato dagli interventi messi in atto da questo Governo e dal ministro Gelmini. Tutti noi che siamo senatori e che coperiamo nei vari territori abbiamo avuto l'occasione di raccogliere le grida d'allarme che vengono dalle scuole, le quali non hanno più risorse neppure per il funzionamento corrente, neppure per garantire la ordinaria amministrazione e vedere

parte integrante dell'ordinamento nazionale dell'istruzione, quindi, costituisce un diritto per quei bambini con le famiglie. Abbiamo sentito tutti la riduzione consistente delle classi di tempo pieno, mentre la domanda delle famiglie aumenta in modo considerevole. Per quanto riguarda riordino della scuola superiore, ci sono preoccupazioni molto, molto gravi, tra cui ad esempio l'accorpamento di classi e, soprattutto, le sparizioni di quelle specializzazioni che danno sbocchi professionali molto importanti per il territorio e per l'occupazione dei ragazzi. Proprio per questo credo che sia indispensabile discutere

per dare chiarimenti relativamente a delle note molto gravi avviate dagli Uffici scolastici regionali, in modo riservato, agli uffici provinciali*...

le priorità da calendarizzare ed anteporre al disegno di legge sulle intercettazioni. Per questo io ne individuo un'altra e la pongo all'attenzione di quest'Aula con riguardo al disegno di legge n. 1464, a mia prima firma, che ha ad oggetto la regolamentazione delle professioni che attualmente non fanno parte di albi, elenchi, od ordini. Si tratta di un mondo di invisibili, di protagonisti del nostro mercato che operano con efficienza che prestano servizi al mondo delle imprese e alle persone e lo fanno con un'alta professionalità, ma non sono riconosciuti. Non essendo riconosciuti non hanno possibilità di operare in un mercato regolamentato e quindi sono assoggettati alla

sulla base di parametri e standard che sono attestati in un sistema di regole, riconosciuto dall'ordinamento giuridico. Per questo è importante riconoscere le associazioni di questi professionisti per far sì poi che in un secondo momento si possa anche garantire loro una tutela previdenziale adeguata perché purtroppo si iscrivono alla gestione separata INPS con costi e contribuzioni troppo alte rispetto alla

Grazie

Riteniamo che la vera responsabilità di quanto accade nel capoluogo dell'isola stia tutta nell'amministrazione guidata dal sindaco Cammarata che spende più energie per incensare il *líder máximo* onorevole Berlusconi anziché per trovare soluzione ai problemi della Al ministro Prestigiacomo vogliamo dare un quadro chiaro della situazione che non ha nei tanto agognati termovalorizzatori la soluzione. Grazie al PD, alla Regione è stata bloccata la vergogna di inceneritori voluti da una commistione chiara tra affari, mafia, cosa nostra e parte della politica, una vergogna costruita sulla illegalità e sulle connivenze. Venga in Aula, ministro Prestigiacomo, e le spiegheremo che le dichiarazioni sulla raccolta differenziata, che qualcuno indica essere già all'80 per cento, sono una bugia: una menzogna che stride con le immagini della Palermo violata, deturpata dalle discariche a cielo aperto. Una gestione scellerata dell'AMIA, l'Azienda per l'igiene ambientale, da parte del responsabile numero 1, il sindaco di Palermo Cammarata, e, a seguire, dei suoi amici, hanno portato al collasso l'azienda, con perdite milionarie, facendo saltare il sistema di raccolta. Venga qui, ministro Prestigiacomo: le spiegheremo come mai l'AMIA ha sperperato le proprie risorse e le faremo capire che non c'è un problema Campania in Sicilia. La questione non sta nel recapito, ma nella raccolta della spazzatura, perché è fallito il sistema di gestione degli ATO. C'è un'emergenza sul sito di Bellolampo, la più grande discarica dell'isola: l'AMIA aveva calcolato in 10.000 tonnellate il percolato, fonte di inquinamento della falda acquifera; un'altra falsità. In verità, le tonnellate sono 100.000. La Regione dovrebbe commissariare il Comune di Palermo; ha deciso invece di anticipare 12 milioni di euro per la bonifica della discarica a causa delle inadempienze del Comune e dell'AMIA stessa. Ministro Prestigiacomo, parleremo dei termovalorizzatori che dovranno realizzarsi con gare vere, nella legalità, contro gli affari, contro cosa nostra, contro i politici corrotti e conniventi. *(Applausi

Signor Presidente, penso sia doveroso prendere la parola sul calendario dei lavori d'Aula che, se approvato, porterà nel giro di pochi giorni alla votazione di una legge che ritengo - come, d'altra parte, moltissimi nel nostro Paese - un colpo durissimo al sistema democratico italiano. Noi sappiamo che dietro a queste norme non c'è la regolamentazione di una modalità investigativa, non c'è lo studio di una disposizione che tuteli la *privacy* e sanzioni il *gossip*, non c'è la disciplina contro gli abusi eventuali di uno strumento investigativo altamente invadente. No. Dietro tutto questo, sappiamo che c'è una visione della giustizia, c'è una cultura politica che ormai sta impregnando anche quest'Aula.

essere modificato e votato, subito. Invece, siamo qui a litigare per evitare che la corruzione vada a finire sui giornali. Strano modo di risolvere i problemi.

grave che presto verrà fatto a quel minimo di Stato di diritto e di cultura del diritto che è rimasta in Italia e a quel massimo, invece, di immagine che ancora continua ad accompagnare il nostro Paese all'interno delle organizzazioni internazionali. Sto parlando, in particolare, del testo unificato o dell'avvio di unificazione di testi relativi all'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale. Come ricorderete, durante la discussione relativa al pacchetto sicurezza, un emendamento presentato, a prima firma dei senatori Poretti e Perduca, e poi sottoscritto da tutti i membri del Gruppo del Partito Democratico, fu posto in votazione, e per soli tre voti non fu provato. emergere di un consenso, che sicuramente andava limato e ulteriormente perfezionato, tutti i senatori del Gruppo Democratico accorparono le loro proposte di legge per l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento, ed emersero

Dicevo che un danno a quel poco di cultura del diritto e a quel tanto di immagine che invece l'Italia ha ancora verrà inferto il 9 giugno prossimo, quando l'Italia sarà chiamata a rispondere in seno al Consiglio dei diritti umani a Ginevra alle raccomandazioni avanzate dall'inizio dell'anno da 52 Paesi. Fra queste, ve ne erano due relative alla tortura. La prima concerne la ratifica del Protocollo aggiuntivo della Convenzione ONU sulla tortura,

mettere magari oggi pomeriggio, domani mattina o sicuramente nei due giorni della settimana prossima, all'ordine del giorno di quest'Aula quel disegno di legge ci farebbe recuperare quel massimo di danno che invece fra due settimane verrà inferto all'Italia insieme alle Nazioni Unite.

In secondo luogo, non le chiederò di cambiare l'ordine del giorno, semplicemente perché mi sarei aspettato, e mi attendo, che il Presidente del Senato, prendendo atto delle dichiarazioni rese dal ministro Alfano uscendo da questo Palazzo («il testo cambierà»), convochi il Ministro, gli chieda conto e ragione delle sue dichiarazioni, cerchi di capire quale sia il testo veritiero sul quale discutere, e lo rimandi in Commissione. Mi aspettavo forse troppo? Forse mi illudo di ritenere fondamentale per la serenità di un percorso legislativo il ruolo del Presidente del Senato, che, in qualità di rappresentante delle istituzioni, deve essere al di sopra delle parti, ma non solo deve essere: deve anche apparire al di sopra delle parti. Si tratta di un ruolo difficile, che richiede equilibrio e senso di responsabilità, come si può evidenziare anche in un semplice comunicato sopra le righe, capace di compromettere sia l'essere che l'apparire del Presidente, un comunicato che recita testualmente: «Il recente clima di sospetti non avvalorati da riscontri probatori da parte della magistratura condiziona e avvelena il clima sociale del Paese». Vale per il Vale per il ministro Bondi, ma anche per chi acquista appartamenti pagati in parte e inconsapevolmente da estranei? Vale anche per chi ha visto confutati requisiti e modalità di elezione? Vale anche per l'evasione IVA di grandi società? Tutti comportamenti che definite eufemisticamente leggeri, superficiali, irresponsabili, e che hanno trovato finalmente un colpevole: la libertà di stampa e la magistratura che utilizza le intercettazioni come strumento di indagine.

Sta a lei, signor Presidente, dimostrare che la politica con la "P" maiuscola ha diritto di cittadinanza in quest'Aula. E si eviti di evocare questioni regolamentari perché torneremmo a quell'essere e a quell'apparire. Essere garante delle regole ed apparire, coadiuvato da cotanti consiglieri che la circondano, un Presidente che per la maggioranza il Regolamento lo si interpreta mentre con l'opposizione lo si attua. No, signor Presidente, sta a lei a due anni dall'avvio della legislatura dimostrare che l'alba di un'latra stagione è iniziata anche per il Senato.

questa settimana alla Camera è stato approvato un decreto che rinvia di tre anni le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero. Si tratta del rinnovo di cariche elettive

affari delle comunità italiane residenti all'estero, uno strumento che sarebbe stato molto utile avere a disposizione in questi due anni, in cui si stanno macellando la rete consolare ed i servizi consolari, si sta uccidendo la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero e si sta procedendo ad una leggera eutanasia dell'immagine dell'Italia nel mondo. Ma prima che mi cada il bavaglio dei tre minuti, nei quali non posso certo parlare dell'importanza di questa Giunta,

per vostra opinione o idea, ma sotto dettato del Governo. Qui si stanno falsando le regole della democrazia e questo è veramente molto grave e pericoloso. Credo che questa mattina le cose si siano mostrate al Paese per come stanno. condanno politicamente questo vostro comportamento di accettare, di vivere e di lavorare sotto dettatura, ma voglio anche esprimere alla maggioranza di voi la mia solidarietà umana nel vedervi in questa legislatura vivere una sofferenza per questa carica,

*(PD)*. Signora Presidente, credo che l'andamento di questa mattinata dimostri come il fatto che in questi mesi il Senato abbia, mesi il Senato abbia, vivacchiato nella discussione per la gran parte di mozioni e di ratifiche di accordi internazionali non fosse legato all'assenza di provvedimenti da esaminare e da approvare, quanto, come avevamo sempre detto, alle difficoltà, alle divisioni e alla paralisi che da subito dopo le elezioni attanagliano questa maggioranza. Voglio portare un altro esempio. Nel corso dell'esame

si impegnarono solennemente di fronte a tutta l'Aula a tornare a breve a relazionare sulle nomine fatte al dipartimento di collaboratori, dipartimento di collaboratori, consulenti e collaudatori e sulle centinaia di assunzioni che hanno trasformato in questi anni il dipartimento in Ministero con portafoglio:e quale portafoglio, i giornali ormai l'hanno specificato. È stato sempre in quella sede, nel corso dell'esame di quel provvedimento, che è emerso come la chiave di volta che ha portato alla mutazione genetica della Protezione civile del nostro Paese sia stata la ormai famosa introduzione dei grandi eventi con il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343. Apprendiamo dalla lettura della stampa che ieri pomeriggio il Consiglio dei Ministri ha licenziato il decreto-legge e

in Parlamento a relazionare su questi due aspetti, perché le novità introdotte e le vicende accadute in questi mesi rendono necessaria una riflessione su quella che dovrà essere in futuro la Protezione civile. Si dovrà sgombrare il campo dai grandi eventi e dalle relative vicende giudiziarie. Io credo che a questo punto, anche per quello che dicono oggi i giornali, sia opportuno che

i giornali di oggi dicono che solo ieri i mercati azionari europei hanno bruciato 113 miliardi ci sono i soldi delle nostre imprese e i soldi delle nostre famiglie. È una situazione molto, molto preoccupante e tutti siamo preoccupati che la crisi finanziaria che sta attraversando l'Europa possa trascinare anche i pur deboli segnali di ripresa economica, che ci sono ma rischiano di essere travolti. Si sta discutendo in questi giorni di provvedimenti in materia. Ieri abbiamo dimostrato grande senso di responsabilità approvando un provvedimento importante per il salvataggio della Grecia e abbiamo dimostrato di assumerci le responsabilità del caso.

Noi abbiamo dimostrato senso di responsabilità, saremmo disposti ad assumerci altre responsabilità e a compiere gesti importanti nei confronti del Paese,

è che, ancora una volta, prevale un'arroganza che noi vorremmo fosse messa da parte: anche di fronte ai nostri gesti di disponibilità a dare a dare segnali costruttivi per il futuro dell'Italia e dell'Europa, da parte della maggioranza c'è un'arroganza che non comprendiamo. Così non si va da nessuna parte e si rischia davvero di fare del male al Paese.

*(PD)*. Signora Presidente, chiedo anch'io una riformulazione del calendario dei lavori dell'Aula della prossima settimana, nonché dell'agenda politica di questo Governo e di quest'Aula. in questo momento la percezione che i cittadini hanno della politica è che essa si occupa troppo di se stessa e troppo poco dei problemi reali del Paese e dei cittadini, dei bisogni e delle attese dei giovani, delle donne e delle famiglie, che ci chiedono di occuparci di loro e ci chiedono di rafforzare e innovare le nostre politiche perché incontrino la loro vita quotidiana. Per queste ragioni ritengo che sia prioritario inserire nel calendario dei lavori di questa autorevole assise, nei prossimi giorni, nella prossima settimana, disegno di legge sulle intercettazioni il disegno di legge n. 784 che, come ricordava anche la collega Blazina, detta misure urgenti a favore della partecipazione delle donne alla vita economica e sociale del nostro Paese. E lo dico perché, se guardiamo alla crisi economica con l'ottica di genere, con l'ottica delle donne, bisogna prendere atto che c'è un *surplus* di gravità nel nostro Paese. La ragione sta nella condizione generale nella quale le donne si trovano a vivere: lavoro scarso e precario, poca carriera, maggiore povertà, carico di cura familiare sempre più accentuato, maggiore esposizione ai licenziamenti, alla cassa integrazione, alla precarietà della condizione di vita. Se non si interviene con questi provvedimenti legislativi efficaci, all'uscita dalla crisi le donne si troveranno sicuramente ancora più povere e ancora più penalizzate nel loro futuro. Questa preoccupazione è fondata, dal momento che le misure che sono state varate fino ad ora segnano davvero un passo indietro: si è cancellata la legge sulle dimissioni in bianco, si sono bloccati i fondi sull'imprenditoria femminile, si sono bloccati gli incentivi alle imprese per assumere donne nel Mezzogiorno, si è messo uno stop al piano di sviluppo degli asili nido previsto dal Governo Prodi, si sono detassati gli straordinari che aumentano il divario salariale tra uomini e donne, penalizzando proprio queste ultime. Ecco perché penso che occorra invece investire sulla risorsa donne per la crescita sociale ed economica del nostro Paese. Sappiamo bene, infatti, che le società nelle quali le donne sono al lavoro sono società più dinamiche e sviluppate. Per queste ragioni chiedo di inserire all'ordine del giorno questo disegno di legge. In sintesi, credo che favorire l'occupazione femminile consentirebbe di rispondere alle esigenze delle donne, di valorizzare una risorsa importante per lo sviluppo economico del nostro Paese e di favorire un efficace mezzo di contrasto alla povertà delle famiglie, rispondendo quindi ad obiettivi di equità, uguaglianza, opportunità ed efficienza economica.

che al massimo entro le prossime due settimane possa essere calendarizzata la discussione del testo unificato del disegno di legge per la riforma degli organismi elettivi di rappresentanza degli italiani all'estero,

1537 e 1990. È urgente e auspicabile che il testo unificato, che porta il nome del suo relatore, senatore Oreste Tofani, venga senza altri indugi licenziato in Commissione per giungere in Aula in via prioritaria rispetto al disegno di legge sulle intercettazioni, di cui peraltro non si conosce ancora la stesura definitiva. La riforma di COMITES e CGIE, il cui rinnovo risulta, incredibilmente e, aggiungerei, illegittimamente, prorogato dal 2009 al 2012, è stata in incubazione ed è attesa da svariati anni; soprattutto, attesa in questo momento di enorme delusione e rabbia delle comunità italiane all'estero per lo stato di abbandono al quale sono costrette da una politica miope di discriminazione e di rinuncia alle iniziative di promozione linguistica e culturale nel mondo e alle iniziative di assistenza sociale per le fasce più deboli dei connazionali espatriati.

*(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, intervengo proponendo anch'io una modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea di lunedì e martedì prossimi, perché ritengo che rispetto al tema delle intercettazioni sia una priorità assoluta il tema della sicurezza alimentare dei cittadini italiani.

per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, che superò la concorrenza di altre città italiane per la sua vocazione territoriale e per la presenza sul suo territorio di punti di eccellenza riconosciuti a livello europeo. Qualche settimana fa il ministro Fazio ha comunicato che questa Agenzia è stata cancellata, perché ritenuta un ente inutile, violando - forse lui non lo sa - le norme europee sulla sicurezza alimentare e danneggiando la sicurezza alimentare di tutti i cittadini italiani.

milioni di euro (peraltro già finanziati), dall'altro si finanzia una scuola europea, il cui costo supera i 46 milioni di euro. Ma si sa che un provvedimento che riguarda il Mezzogiorno è un carrozzone e ciò che supera la linea gotica» è un atto dovuto! a tutti i colleghi che, senza le olive meridionali, l'Italia sarebbe senza olio, senza i pomodori del Sud non potremmo condire la pasta e, senza il nostro grano, non avremmo ovviamente la splendida pasta italiana. Vivaddio, in questo Paese c'è qualcosa che ci unisce!

che dobbiamo fare questi sacrifici, ma c'è una speranza, e manca la capacità di chi dirige il Paese di offrire un indirizzo circa i mutamenti che sono necessari per recuperare la capacità competitiva del sistema Italia, senza la quale le misure che oggi prendiamo non solo saranno sostanzialmente inutili, ma rischiano di essere addirittura controproducenti. Non dobbiamo dimenticare l'esempio del 1937, che pochi ricordano: in quell'anno, errori di politica fiscale del Governo americano, clamorosamente in contraddizione con gli orientamenti che erano prima prevalsi dopo l'esplosione della crisi del 1929, 1929, finirono per determinare un rimbalzo all'indietro del contesto della crisi, da cui si poté uscire soltanto alla fine della Seconda guerra mondiale. bisogno di riforme strutturali che forniscano un robusto contesto politico alle misure immediate di risanamento, che pure sono necessarie e debbono essere prese. Colleghi della maggioranza e del Governo, qualche scelta su questo versante? Vi propongo allora di iscrivere all'ordine del giorno, al posto del provvedimento sulle intercettazioni, il disegno di legge n. 2102, di cui mi onoro di essere primo firmatario, con il quale si propone una drastica riduzione delle aliquote di prelievo IRPEF sui redditi da lavoro dipendente delle donne, cioè di quella che rappresenta oggi probabilmente...